finestra"). In data 14 novembre 2006, è stato presentato il seguente disegno di legge: *dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale:* «Conversione in legge del decreto-legge 13 novembre 2006, n. 279, recante disposizioni urgenti in materia di previdenza

ma pure i colleghi dell'Assemblea, visto che è un argomento in discussione anche in Aula, che la 1a Commissione affari costituzionali, da me presieduta, ieri era pronta a esprimere il suo parere

da parte del Governo di essere presente quando le Commissioni sono riunite in sede consultiva, ho ritenuto comunque, vista la particolare delicatezza e complessità delle questioni sollevate in Commissione affari costituzionali, che la Commissione stessa non potesse deliberare in assenza delle risposte richieste dal Governo. aggiornato la seduta ad oggi pomeriggio e ho personalmente richiesto e raccomandato al Governo di essere presente per fornire le risposte che erano state richieste, purtroppo la Commissione non ha potuto deliberare perché anche oggi pomeriggio il Governo non era presente: mentre era presente durante la trattazione di altri punti all'ordine del giorno, durante la trattazione Ripeto: non c'è uno stretto obbligo regolamentare ma, signor Presidente, apprezzerà il fatto che si tratta di una questione particolarmente delicata, per cui la Commissione in modo unanime ha condiviso la mia scelta. Non potevo non far osservare quanto accaduto e chiedo alla Presidenza del Senato di manifestare il profondo rammarico

Siamo di fronte a un decreto-legge che il Governo considera così importante da averlo inserito come provvedimento collegato al disegno di legge finanziaria, indispensabile quindi ai fini del completamento della manovra di politica economica e finanziaria del Paese. Già nella scorsa settimana, in 1ª Commissione affari costituzionali, nel discutere i presupposti di necessità e di urgenza, un rappresentante del Governo, da me personalmente interpellato nel corso del dibattito per avere l'opinione del Governo, aveva risposto che ad avviso dell'Esecutivo esistevano i presupposti di necessità e urgenza. Siamo a un livello tale che una lezione di educazione civica agli studenti delle scuole elementari probabilmente sarebbe più congrua. Perché faccio questo ragionamento, signor Presidente? Perché siamo di fronte a un decreto‑legge. Il decreto‑legge è di regola vietato dall'articolo 77 della Costituzione, al secondo comma, stabilisce che in determinate circostanze il Governo può emanarlo assumendosene la responsabilità. Quando un Governo deve assumersi, ai sensi della Costituzione, la responsabilità di un provvedimento, ha l'obbligo di venire in Commissione, al di là dei Regolamenti, a motivare, soprattutto quando la Commissione lo richiede. Viviamo in un sistema di democrazia parlamentare, rispetto al quale il rapporto tra i diversi poteri dello Stato o si realizza in Parlamento o non si realizza. Non capisco come il Governo possa ritenere di potere andare avanti senza presentarsi in Commissione, quantomeno per dire che non intende esprimere la propria opinione o per rimettersi alla volontà della Commissione. La

per ciò che il Parlamento rappresenta come potere legislativo nel Paese e per i rapporti del Parlamento con il Governo. Nella mia lunga esperienza parlamentare non si è mai verificata l'ipotesi di assenza del Governo su decreti-legge nel momento in cui bisognava discutere della loro costituzionalità. Vogliamo introdurre anche questo tipo di costume? Presidente,

aggiungendo un elemento che serva da valutazione anche per la Presidenza del Senato. L'unica difformità che ho nei riguardi dell'opinione espressa dal collega Bianco è che non ci sia, secondo la sua autorevole opinione, obbligo del Governo ad essere presente in sede consultiva. Stiamo parlando di un decreto-legge; sui profili di costituzionalità credo che l'obbligo sia in sé, ma quello che conta è la sostanza, più che la forma. E la sostanza - lo voglio ricordare all'Aula, signor la differenza sul parere, almeno limitato a quattro commi del decreto-legge, era che da parte della maggioranza bastava un'osservazione, da parte della minoranza serviva una condizione. Questa è la questione. Ma tutta la Commissione (in quel parere non votato perché non c'era la presenza del Governo) era concorde nell'avere quantomeno dubbi su quattro commi del decreto collegato alla finanziaria. Allora, signor Presidente, qual è il problema che si pone? Noi saremo impossibilitati ad intervenire, sia la minoranza che la maggioranza, almeno su tale questione a causa dell'interpretazione che si è data ieri al Regolamento con la votazione a norma dell'articolo 102, per cui si è deciso che l'Assemblea prende tutto o niente per discutere, e si è evitato a colleghi di maggioranza e di minoranza di convergere su una questione. In secondo luogo, come lei mi insegna (il Regolamento è

- consentire che si possa votare almeno una pregiudiziale su quattro commi. Forse su questo faremmo scuola per il futuro, perché se un'Assemblea

che ho qualche dubbio che la discussione di merito si concluda con la fiducia, credo che rischieremo di portarci appresso una norma incostituzionale, sulla quale noi abbiamo espresso certezze sulla incostituzionalità e la maggioranza dubbi sulla costituzionalità, con il risultato - lo ripeto - che ce la portiamo appresso così com'è, rischiando di fare dei danni.

a parte rispetto alle pregiudiziali. È una questione che riguarderà la giornata di domani; è chiaro che la questione non la possiamo porre in forza di un Regolamento, ma la dobbiamo porre in forza della saggezza che deve guidare un'Aula nell'evitare che si approvino norme che possono essere inficiate da incostituzionalità.

al mio dovere di dare un piccolo contributo al dibattito. Il provvedimento in discussione è assai complesso e l'eterogeneità delle disposizioni contenute nei 48 articoli di cui si compone è giustificata dalla funzione stessa del decreto‑legge in questione, in quanto esse concorrono alla manovra di finanza pubblica per il prossimo anno. Il provvedimento, infatti, si presenta, in modo unitario e coerente, come un intervento complessivo, orientato a dettare norme relative agli aspetti fiscali e di finanza pubblica, quale integrazione e presupposto indispensabili della manovra di bilancio. Perciò, la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, sta nella straordinaria necessità...

chiudo qui il mio intervento, come se non fosse stato svolto.

Ora lei dice: ci auguriamo che domani il Governo sia presente. Stia certo che il Governo sarà presente al gran completo, perlomeno la sua rappresentanza senatoriale. Noi abbiamo la necessità di sapere dal Governo se le questioni poste,

si stralcino quelle norme e se il Governo sia consapevole del rischio di scontro di fronte alla Corte costituzionale. Sono, infatti, messi in discussione i diritti di cittadini privati che hanno lavorato con lo Stato e di dipendenti pubblici che non vengono risarciti.

italiana. Stiamo parlando di un decreto per il quale siamo disponibili anche noi a lavorare giorno e notte, come dimostra la battaglia parlamentare. Non è tollerabile che non si risponda a una questione di costituzionalità che è ormai riconosciuta da tutti.

Il Resoconto stenografico di oggi sarà un motivo in più per far riflettere sull'esame delle pregiudiziali di costituzionalità. Quindi, rinnovo l'invito alla prudenza nell'affrontare domani tale problema, perché credo che si abbia il diritto di esaminare separatamente la questione dei commi - su cui almeno c'è stata una condivisione di dubbi - dal 159 al 162. Grazie, senatore Storace. La Presidenza, anche perché ha vissuto personalmente entrambi gli episodi, non può che condividere quanto indicato dal presidente Bianco e dai colleghi che si sono associati. Esprimo, proprio a nome della Presidenza, un rammarico, perché se manca un obbligo regolamentare, perché c'è solo in sede referente, credo che su un decreto‑legge collegato alla legge finanziaria, su precisa richiesta del Presidente della Commissione nel giorno antecedente il voto, sarebbe stato estremamente opportuno venire a fornire quelle motivazioni che sono state introdotte ora ma in una sede assolutamente inopportuna. Mi auguro che domani, quando discuteremo pregiudiziali e sospensive, ci sarà l'occasione per verificare se tali requisiti non siano urgenti e necessari solo perché sono urgenti e necessari, come talvolta sembra di capire. Pertanto, esprimerò il mio rammarico al ministro Chiti,

nodo centrale per le questioni della democrazia. Uno dei punti centrali della vertenza sul contratto dei giornalisti è proprio la condizione di precarietà di circa 30.000 lavoratori del settore. Ritengo utile, proprio per dare consequenzialità al richiamo così autorevole del Presidente della Repubblica, chiedere al Ministro del lavoro, che per il Governo segue la possibilità della ripresa di un tavolo di trattativa tra giornalisti e editori, di riferire in Parlamento sullo

Credo sia rilevante per il Paese e per il Senato, anche in funzione della discussione che a breve si farà sui contenuti della finanziaria e del decreto fiscale che, appunto, parla

mi associo a quanto testé detto dal collega, sottolineando anche un aspetto accessorio, ma molto importante di quella vertenza.

il senatore Malan. La Presidenza inviterà il Ministro del lavoro a venire a riferire in Aula. Auguriamoci che la vertenza si risolva quanto prima, in modo che non si ponga neppure il tipo di problema segnalato dal senatore Malan.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento che stiamo per votare ha il grande pregio di essere un provvedimento per i giovani e per il futuro del Paese. Le migliorie che il Governo e il Parlamento hanno voluto apportare alla precedente regolamentazione dell'esame di Stato sono efficaci e di grande spessore, in quanto richiedono un impegno maggiore da parte degli studenti e, soprattutto, una loro responsabilizzazione che consiste non solo nel conseguire risultati scolastici di buon livello, ma anche nel mantenere nel tempo un rendimento qualitativamente elevato. A tale proposito è significativa l'importanza che il presente provvedimento attribuisce alla verifica dei risultati conseguiti dagli studenti per tutta la durata del percorso scolastico richiedendo, come requisito necessario per l'ammissione all'esame di Stato, non solo una valutazione positiva in sede di scrutinio finale, ma anche il recupero dei debiti formativi eventualmente contratti negli anni scolastici precedenti. Inoltre, per conferire ulteriore serietà alle prove e maggior valore al titolo di studio che negli ultimi anni è andato svilendosi, perdendo prestigio in ambito europeo, la volontà del Governo di contrastare i cosiddetti diplomifìci ha stabilito regole rigorose per gli studenti che sono ammessi all'abbreviazione del corso di studi, al fine di rendere qualificanti ed autentici i percorsi dell'eccellenza. A tal fine vengono, infatti, presi in considerazione i punteggi ottenuti in tutte le materie, non solo durante la penultima classe frequentata, ma anche nei due anni antecedenti il penultimo. Per essere ammessi, i candidati esterni devono superare un esame preliminare e possono sostenere l'esame di Stato presso istituzioni scolastiche statali o paritarie che hanno sede nel Comune di residenza. Tale passaggio è molto importante in quanto afferma l'appartenenza a pieno titolo delle scuole paritarie al sistema pubblico di istruzione, ma altresì stabilisce per tutti il rispetto di identiche regole in merito all'ammissione degli alunni all'esame, alla scelta delle sedi d'esame e, soprattutto, alle modalità di svolgimento delle prove. Possono essere ammessi a sostenere l'esame di Stato anche candidati esterni appartenenti a Paesi dell'Unione Europea e questa novità non solo promuove un processo di integrazione con gli altri Stati membri, ma istituisce, insieme all'adozione di criteri e modalità di valutazione coerenti con quelli applicati a livello internazionale, la comparabilità dei titoli conseguiti. Per quanto riguarda il contenuto dell'esame di Stato, si è posto l'accento sulla verifica dei risultati conseguiti nell'ultimo anno del corso di studi, prendendo in esame tre prove scritte ed un colloquio. I testi della prima e della seconda prova sono scelti dal Ministro, mentre la terza prova, scelta dalla commissione d'esame, diventa espressione dell'autonomia scolastica. La valutazione che ne consegue terrà conto degli obiettivi e dei campi di applicazione specifici di ciascun indirizzo, nonché di nozioni di cultura generale e delle personali capacità critiche dei candidati, e sarà espressione del livello di conoscenza e capacità raggiunto dagli studenti alla fine del percorso scolastico. Altri elementi innovativi sono costituiti dalla possibilità, da parte della commissione d'esame, di attribuire la lode in caso di eccellenza, nonché dalla composizione della commissione stessa, che sarà costituita da non più di sei commissari per metà interni e per l'altra metà esterni, più il presidente, ovviamente esterno. Infine, la novità di vero rilievo strategico è costituita dalla delega al Governo ad adottare decreti legislativi per promuovere percorsi di orientamento universitario, di formazione artistica e musicale, di indirizzo verso istituti che garantiscano una specializzazione di livello tecnico superiore e, in ogni caso, percorsi che guidino i ragazzi verso il mondo del lavoro. Il nostro compito è ora quello di approvare con urgenza questo provvedimento per consentire alle istituzioni scolastiche di prendere immediato contatto con la nuova disciplina, non solo per il bene dei ragazzi, ma per quello della scuola italiana nella sua interezza. Ed è nell'interesse per questo percorso che accompagna i ragazzi dalla scuola dell'obbligo, dagli anni difficili dell'adolescenza e della formazione a quelli della specializzazione universitaria, dell'approfondimento tecnologico, artistico e professionale che lo Stato manifesta il suo vero e profondo impegno nei confronti delle nuove generazioni,

Onorevoli colleghi, anche oggi dobbiamo purtroppo manifestare per l'ennesima volta un parere contrario ad un disegno di legge presentato da questo Governo. legge in questione, infatti, sul solco di molti altri provvedimenti già passati in quest'Aula, non apporta nessuna reale o significativa novità, o non si propone alcuna reale riforma per risolvere le tante, lamentate criticità della scuola italiana. Ancora una volta, quindi, dobbiamo amaramente constatare come l'intento palese e manifestato sia quello di smantellare, pezzo per pezzo, tutte le maggiori riforme attuate dal precedente Governo, senza tuttavia riuscire, contemporaneamente, ad individuare alcuna reale tendenza riformatrice, volta a dare soluzioni alle mille problematiche sollevate continuamente e costantemente negli anni passati sull'operato del Governo Berlusconi. Da un lato, si proclama di voler mirare ad una scuola più efficiente, funzionale e adatta ad inserire i nostri giovani nel duro mondo della competizione lavorativa, che ha oramai confini europei, ma dall'altro, nel disegno di legge finanziaria, attualmente in discussione alla Camera, si penalizza fortemente tutto il settore dell'istruzione e in particolare quello universitario. I soldi sono pochi

in questo disegno di legge, di reintrodurre la figura del membro esterno nella commissione esaminatrice, che porterà inevitabilmente con sé maggiori costi. Di certo, non sarà questa figura a poter garantire, in maniera efficace, un esame rigoroso e selettivo. Le previsioni di questo disegno sono sicuramente troppo deboli e prive di una reale capacità di incidere sull'attuale assetto scolastico o anche solo sul fondamentale passaggio conclusivo, costituito dall'esame di maturità. Inoltre, si può facilmente notare come molti dei punti qui in approvazione oggi altro non siano che previsioni già contenute nella riforma Moratti, oggetto di molteplici critiche. Pensiamo, ad esempio, al necessario superamento dei debiti per l'accesso all'esame stesso. Molti dubbi sollevano, alcune previsioni, come ad esempio quella contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, relativa alla possibilità, delegata al Governo, di poter introdurre una limitazione all'accesso all'istruzione universitaria sulla base dei risultati scolastici precedenti, contrastando questa, prima di tutto, con il principio del diritto allo studio e, successivamente, con l'autonomia degli atenei. Oppure, la previsione contenuta nell'articolo 1, comma 6, che consente agli alunni, non appartenenti a Paesi dell'Unione Europea che non abbiano frequentato l'ultimo anno di istruzione secondaria superiore, di poter sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni, generando così una ingiusta disparità di trattamento con i nostri ragazzi. La nostra non è una critica fine a sé stessa, abbiamo a cuore il futuro delle nuove generazioni, la linfa del nostro Paese, e siamo aperti ad dialogo costruttivo; ma essenziale è sicuramente l'individuazione di precise priorità da perseguire. I problemi sono molti, anzi moltissimi, e non ci sembra corretto perdere tempo, energie, denaro pubblico su dettagli poco costruttivi o senza reale capacità incisiva. La riforma Moratti, con tutti i suoi pregi, ma anche con tutti i difetti che può avere, ha avuto il merito di mirare a una riforma strutturale e d'insieme del settore scolastico, individuandone le criticità e proponendo delle soluzioni. Si sa, nulla è perfetto e tutto è perfettibile, ma lo sforzo è stato enorme e gli intenti sicuramente lodevoli. Ma possiamo dire altrettanto di queste proposte? Sicuramente anch'esse propongono punti di interesse, ma evidentemente non presentano la medesima visione di insieme, né individuano soluzioni incisive. Da un lato, infatti, si riconosce il valore e si riafferma la dignità dell'esame conclusivo della scuola superiore, consacrato come principio dalla nostra Carta costituzionale, ma, dall'altro, la sua estrapolazione da un complesso di riforma più organico contraddice questo intento, peraltro, di per sé stesso, condivisibile. Tutto ciò ci porta a dover ribadire con forza il nostro no a tale intervento che nulla aggiunge, ma che conferma, al contrario, solo una precisa volontà di smantellare, pezzo per pezzo, quanto già fatto, senza minimamente pensare a cosa a cosa ciò porterà di realmente utile per il nostro Paese. La congiuntura economica grava sul nostro Paese e il Governo non sta fornendo risposte adeguate o lungimiranti; questo disegno di legge ne è solo un piccolo esempio.

Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il Gruppo Per le Autonomie condivide gli obiettivi della riforma degli esami per la scuola secondaria superiore. Con questa riforma, infatti, si risponde a un'esigenza sociale, sentita non solo dai docenti, dalle imprese e dall'università, ma soprattutto dagli stessi ragazzi, che rappresentano il futuro del nostro Paese. L'esame di Stato - la «maturità» - riacquista di serietà, facendo emergereil profilo di una scuola solida nelle basi culturali, aperta, che riconosce il merito, valorizza i talenti ed è sensibile ai risultati. Tutto ciò va a vantaggio degli studenti e rende la nostra scuola più europea, con l'obiettivo di rafforzare l'impegno dell'Italia verso sé stessa e verso il proprio domani. Questa è la terza legislatura in cui il Parlamento si occupa e cerca di affrontare la questione degli esami di Stato. Il testo su cui siamo chiamati a votare, predisposto dal Governo e modificato, vorrei anche dire migliorato, in 7a Commissione, è stato arricchito da numerose audizioni ed è anche il risultato di un confronto costruttivo tra maggioranza ed opposizione. Devo dire che questo clima, di cui mi è stato riferito, della 7a Commissione purtroppo poi non si è risentito in Aula, ovviamente per motivi politici palesi. L'esame di Stato segna, per ciascun adolescente, il passaggio all'età adulta, ad una nuova fase di studio e di lavoro. È per questo che la riforma degli esami di Stato è un atto doveroso, per migliorare e qualificare al massimo la prova di maturità. Gli studenti, infatti, hanno diritto di veder valorizzata la propria esperienza scolastica e di veder riconosciuti i risultati acquisiti. Come evidenziato dalla relatrice, senatrice Albertina Soliani, che ringrazio per il suo lavoro, tre sono i punti qualificanti il provvedimento in questione. la natura pubblica dell'esame, il contrasto delle cosiddette fabbriche dei diplomi (che troppo facilmente, anche su pagamento, fornivano questi diplomi), la serietà delle prove di maturità e dell'impianto ed il valore del titolo di studio, che con questo sarà valorizzato. la responsabilizzazione degli studenti e delle istituzioni scolastiche, anche in ordine alla verifica dei risultati, nella valorizzazione delle autonomie scolastiche. l'orientamento e il raccordo con l'università, gli istituti tecnici e musicali, le professioni del lavoro. Per contribuire al miglioramento del testo, anche il Gruppo per le Autonomie, che ho l'onore di presiedere, aveva presentato una serie di emendamenti. Salutiamo pertanto con favore l'accoglimento del nostro emendamento teso a salvaguardare lo svolgimento dell'esame di maturità nella Valle d'Aosta, in merito ad una quarta prova scritta in lingua francese. Ribadiamo anche la specialità dell'esame di Stato nella Provincia autonomia di Bolzano; è già previsto dalla legge costituzionale e da quella ordinaria che l'insegnamento e l'esame si svolgano nella lingua dell'alunno e, per la scuola tedesca, si svolgano appunto in lingua tedesca. Il disegno di legge correttamente prevede, inoltre, che la prima prova scritta, intesa ad accertare la padronanza della lingua, si svolga in lingua italiana o nella lingua in cui è stato svolto l'insegnamento, tenendo conto praticamente della protezione delle minoranze linguistiche; di questo prendiamo atto con soddisfazione. Restano comunque dei punti aperti, su cui, come Gruppo per le Autonomie, avevamo chiesto un intervento correttivo. Nello specifico, avevamo chiesto di aggiungere all'articolo 1 che, nei confronti degli alunni i quali, al termine dell'ultimo anno di corso, presentino un'insufficienza non grave in non più di due discipline, comunque non tale da determinare una carenza grave nella preparazione complessiva, si applichi una procedura più approfondita. Il consiglio di classe dovrebbe procedere, ai fini della valutazione positiva o negativa complessiva degli stessi, in sede di scrutinio finale, sulla base di parametri valutativi stabiliti preventivamente, ad una valutazione che tenga conto della possibilità o meno dell'alunno di superare l'esame di Stato. Inoltre, era nostro intento far inserire, sempre all'articolo 1, che, ai fini dell'ammissione all'esame di Stato, la promozione degli alunni all'ultimo anno di corso equivale al saldo di tutti i debiti formativi contratti negli anni scolastici precedenti, ad eccezione del penultimo anno in corso. Riguardo ai presidenti delle commissioni d'esame, avevamo chiesto che questo ruolo potesse essere svolto anche dai dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti di istruzione secondaria superiore paritari.

In ultimo, il Gruppo Per le Autonomie aveva proposto che, qualora il colloquio della prova di esame riguardi argomenti attinenti alle lingue straniere, lo stesso può essere svolto nella lingua straniera. con la versione della legge la quale dice che l'esame si svolge nella lingua dell'alunno, potrebbe essere precluso; ciò mi sembra ovvio, però spero che nelle direttive sia chiarito. Abbiamo deciso di ritirare questi ultimi emendamenti dopo le assicurazioni forniteci dalla relatrice Albertina Soliani e dalla vice ministro Mariangela Bastico, che ringraziamo, che ci hanno confermato la piena disponibilità del Governo a riprendere le nostre proposte e a concordare, per quanto riguarda le nostre specialità, con il nostro Gruppo le direttive che verranno emanate alle scuole per l'applicazione della futura legge. Grazie per questo. Ci auguriamo pertanto che il Ministro provveda a recepire la sostanza delle nostre proposte ai fini della piena valorizzazione dell'autonomia delle Regioni e Province a Statuto speciale. Egregio signor Presidente, onorevoli colleghi, concludo annunciando il voto favorevole del Gruppo Per le Autonomie. Signor Presidente, signor Vice ministro, onorevoli colleghi, il testo che abbiamo di fronte è un testo equilibrato, e credo che proprio il suo elaborato riuscirà in quello che era l'obiettivo primario della proposta normativa, cioè ridare serietà e rigore all'esame di Stato come unico argine alla tentazione di eliminare il valore legale dei titoli di studio. La commissione mista e la reintroduzione dell'ammissione all'esame sono elementi importanti della riforma, una riforma che mi auguro possa essere oggi approvata da quest'Aula e, presto o poi, dall'altro ramo del Parlamento, per dare certezze agli insegnanti e agli studenti che stanno svolgendo l'anno scolastico. Ma l'elemento sul quale ritengo utile soffermarmi è quello che, se oggi è solo accennato con la delega contenuta nel testo nei confronti del Governo, può diventare un elemento qualificante della scuola che vogliamo costruire: con l'orientamento all'università si avvia un processo fondamentale che è quello di fare della scuola il centro di un sistema territoriale di formazione lungo il corso della vita. Ho molto insistito sull'orientamento al lavoro durante i lavori in 7a Commissione, sulla possibilità di costruire un percorso d'ingresso nel mercato del lavoro con piena dignità da parte dei nostri studenti proprio perché sono convinta che oggi solo la scuola possa essere quel motore capace di riorientare verso la società della conoscenza il nostro tessuto produttivo e i soggetti che compongono il territorio. Sono certa che, se oggi iniziamo questo percorso con l'orientamento universitario, il Governo e il Parlamento avranno modo di affrontare anche questo impegnativo capitolo. L'insieme composto dal provvedimento che stiamo esaminando e che fra poco voteremo e da alcune proposte contenute nella finanziaria, come i centri di educazione degli adulti e l'innalzamento dell'obbligo scolastico a sedici anni, possono essere la strada per raggiungere questo obiettivo, quello della formazione lungo il corso della vita, una formazione moderna e orientata all'autonomia dei cittadini. Ma, lo ripeto, solo la scuola può essere il promotore di questo impegnativo percorso. E puntualizzo: solo la scuola pubblica. Nella nostra discussione è ripetutamente echeggiata la questione della legge di parità, che definisce la composizione del servizio scolastico pubblico. Essa è stata addirittura al centro della questione pregiudiziale posta dall'opposizione all'inizio dei nostri lavori ed è ritornata spesso negli interventi di stamattina. Secondo me non occorre equivocare sulle parole: restano delle profonde differenze, che la stessa legge sulla parità conferma, tra scuole statali e scuole paritarie. Non si può affermare che, perché ai sensi della legge di parità entrambe concorrono a definire il servizio pubblico, sono la stessa cosa: scuole statali e scuole paritarie non sono la stessa cosa, lo dice la legge sulla parità. Per esempio, la proposta che anche i docenti della scuola paritaria potessero essere membri esterni nella scuola statale avrebbe introdotto una premialità inaccettabile per tipologie di lavoratori che, se concorrono allo stesso servizio pubblico, hanno una differenza di fondo: gli uni dipendono dallo Stato, gli altri da amministrazioni di altra natura. Ed è proprio per cogliere le differenze, con puntualità, che questa norma introduce passaggi importanti contro i «diplomifici», come la commissione mista, l'esame preliminare, un massimo di trentacinque candidati per commissione. Ma per raggiungere questo obiettivo è necessario un impegno continuativo, e sono certa che il Ministero saprà dimostrare questo impegno. Se non saremo in grado di eliminare i «diplomifici» ogni nostro sforzo per riformare l'esame sarà stato vano. L'esistenza di strutture dove, con quattro soldi, si può letteralmente comprare il diploma svilisce il ruolo della scuola e l'impegno dei docenti nel costruire tutti i giorni una scuola rigorosa ed equa, ma soprattutto incide pesantemente sul nostro sistema produttivo e non consente una seria politica per valorizzare le eccellenze. Oggi, con questo atto dovremmo finalmente aver posto fine a questa piaga, in crescita costante negli ultimi anni, e costruito un percorso serio per il rilascio del diploma. Spero che abbiamo costruito un lavoro sufficientemente condiviso da durare nel tempo e che non si riveli, come preconizzava nel dibattito un collega di Alleanza Nazionale, una norma transitoria: gli esami di maturità - è già stato ricordato - vennero introdotti per via sperimentale nel 1967 e riformati e resi stabili nel 1997, trent'anni dopo. Da allora ad oggi, in soli dieci anni, questa è la terza riforma a cui assistiamo. Questa della quale discutiamo era certo indispensabile, come dimostrato dal fatto che anche le opposizioni, proponendo loro testi di riforma, abbiano preso atto che la riforma precedente era lacunosa. Ma spero che la scuola non debba affrontare ogni tre anni una riforma degli esami. L'idea che ad ogni cambio di maggioranza cambino le regole sarebbe perniciosa per la scuola. Oggi spero che si sia costruita una riforma capace di durare nel tempo, e capace anche di essere quel punto fisso su cui costruire nuove e importanti politiche per la scuola. Penso al passaggio che abbiamo di fronte, particolarmente importante, cioè la certificazione delle competenze reali degli allievi, soprattutto rispetto al mondo del lavoro. L'esame di Stato avente valore legale con il punteggio definisce un livello quantitativo di competenze, ma non ne definisce la qualità: definisce quanto l'allievo sappia, non cosa sappia. Avremo modo di discutere di una scuola flessibile, capace di dare a ciascuno secondo il bisogno proprio del singolo allievo, e capace di certificare il percorso di ciascuno, come già molte Regioni sperimentano con i libretti formativi. Per questo abbiamo fortemente voluto che l'orientamento riguardasse anche il mondo del lavoro e che ci fosse un'attenzione privilegiata per le materie tecnico-scientifiche: perché vogliamo costruire una scuola che sia il punto di partenza per la formazione nel corso della vita di ogni cittadino. Oggi, dopo l'approvazione del provvedimento al nostro esame, tutte queste politiche possono finalmente essere attuate, e sono politiche necessarie, perché permetteranno alla scuola di essere più efficiente e flessibile, agli studenti di essere più competenti, al sistema produttivo di essere più competitivo.

cose sono già state dette nel corso della discussione. Mi vengono in mente tre aggettivi: inutile, intempestivo, inopportuno. È il giudizio a caldo, immediato, nei confronti di questo provvedimento. Inutile, perché

viene imposto nel breve periodo; l'anno è in corso: chi l'anno scorso è stato promosso con tre debiti formativi

vero determinato dal titolo di Stato, da quella dichiarazione che lo Stato fa nei confronti di quel ragazzo, di quel cittadino. Pertanto all'alto valore del titolo di Stato vogliamo che corrisponda veramente - ne siamo tutti convinti - il vero della formazione dei nostri ragazzi. Si perderà in autonomia, perché le tre prove arriveranno tutte dall'alto. È stato fatto il tentativo, vi abbiamo contribuito anche noi e ne siamo in in parte soddisfatti, ma sappiamo che non sarà così: le tre prove d'esame arriveranno dal centro, dall'alto, con un'impostazione

Provvedimento inutile in tal senso ed intempestivo, perché arriva a metà di un anno scolastico, di un anno formativo. Le famiglie non vanno prese in giro, vanno seguite.

hanno bisogno di regole chiare e certe su cui adattare la loro libertà, la loro fantasia e la loro creatività. Cambiare le regole a questo punto significa non rispettarli, significa non rendere loro un buon servizio e non rendere un buon servizio alla scuola. anche inopportuna, perché diventa dispendiosa e quell'inserimento dei commissari esterni si traduce in una mancanza di fiducia nei confronti degli insegnanti che hanno formato quei ragazzi. Di fatto il

punte del 30 per cento, e cosa fa il Governo? Niente, pensa alla fine e pensa all'inizio. Innalzare l'obbligo scolastico non significa combattere la dispersione scolastica, perché dalla terza media alla prima classe delle scuole superiori la dispersione scolastica non dico che non esista ma è ridotta ai minimi termini (3 o 4

dal punto di vista economico, che non ce la faranno a sostenerli o li sosterranno con molta difficoltà. Si sono salvati forse alcuni corsi sperimentali nati in alcune Regioni, speriamo almeno quelli, anche se non ne ancora abbiamo la certezza perché la finanziaria è ancora in fase di definizione.

ciò che esso non fa. Per dare solamente una parvenza di aver fatto qualcosa in realtà non si è fatto proprio niente. Non si è fatto niente dove bisognava fare qualcosa e si è invece fatto qualcosa dove non bisognava farlo, dove non bisognava toccare, dove nessuno sentiva l'esigenza di fare Ma c'è ancora un'altra situazione di cui voglio parlare. Sono andato a vedere tutti i cambiamenti che stanno per essere introdotti. Questo Ministro aveva annunciato che non voleva dare il proprio nome ad una riforma. In realtà, questa riforma la sta già attuando, perché sono oltre sono oltre venti i provvedimenti attuativi che verranno delegati direttamente al Ministro e che riguarderanno la scuola. Sono venti provvedimenti, venti passaggi importantissimi che costituiscono una riforma.

È la prova di ciò che stiamo dicendo, non solo di un cattivo Governo e di una cattiva amministrazione del nostro sistema, ma della volontà

deve necessariamente passare attraverso il confronto di tutti, maggioranza e minoranza, perché la scuola - e ciò è stato detto dal Ministro e da molti di voi in quest'Aula - è di tutti; e, se è di tutti, tutti devono essere ascoltati, tutti devono partecipare e non essere trascurati, lasciando tutto nelle mani di un Ministro solo.

ancora l'esame degli emendamenti in Aula ha confermato quanto già ci siamo detti in sede di dibattito generale: questo disegno di legge era già blindato fin dal suo nascere, come quasi tutte le proposte fatte dal centro-sinistra in Senato, fatte salve poche lodevoli eccezioni che abbiamo avuto modo di apprezzare come Gruppo UDC. Perché non possiamo esser d'accordo con questo disegno di legge? Perché riteniamo che non si può cominciare a ragionare dal tetto della casa per capire quale casa si deve costruire o ristrutturare o semplicemente riammodernare. Certamente suggestiva la citazione che la relatrice Soliani ha fatto di Benedetto Croce, ma non per questo convincente. Croce forse parlava di una scuola che aveva una sua struttura e una sua tradizione ben definita e comunque in un tempo che non consente raffronti sociali di alcun genere. Far partire una revisione e una verifica cominciando dall'esame di maturità, facendolo diventare una sorta di stella cometa che guidi e illumini ogni cosa, quando questo è evidentemente alla fine di un processo, mi sembra eccessivo, come eccessiva è l'importanza che allo stesso esame di maturità si vuole attribuire. Ben altre dovrebbero essere le considerazioni che ci muovono intorno alla scuola, con la capacità di vedere innanzitutto una società che si muove non solo rapidamente, ma anche molto più liberamente di un tempo. È singolare il fatto che la maggioranza, attualmente al Governo, avverta tutti i cambiamenti in campo etico e sociale, magari forzandone finanche la reale necessità, come nel caso dei PACS, ma non sia capace di vedere come sia cresciuta la voglia e la facoltà di gestire nuovi spazi di libertà da parte dei cittadini, per esempio in campo educativo e scolastico, con l'evidente volontà di non essere più e solo ancorati all'unica scuola di Stato, intorno alla quale dovrebbe concentrarsi secondo voi tutto il sistema formativo italiano. Questa riforma dell'esame di maturità ne è una spia evidente e per noi, moderati e cattolici democratici, anche abbastanza preoccupante. Non sto facendo illazioni o supposizioni forzate, sto a quello che ha affermato la stessa relatrice nella presentazione del disegno di legge. Ha detto: «Tre i punti qualificanti del presente provvedimento: il primo è la natura pubblica dell'esame e il contrasto dei «diplomifici», la serietà delle prove e dell'impianto, il valore del titolo di studio». La natura pubblica dell'esame, quindi, sta a contrastare il «diplomificio», che - è già stato affermato - viene identificato soprattutto nella scuola privata, da sempre rea di poca serietà nella prova e nell'impianto. Traspare, neanche troppo velata, la vecchia convinzione che tutto il bene è nel pubblico e tutto il male, o quasi, nei privati. Non voglio cadere nell'errore opposto, ma credo che questa cultura non ci porterà lontani: in questa mentalità è assente il rischio, l'innovazione, lo spirito creativo, la responsabilità della gestione della cosa pubblica lasciata ad altri che non sia lo Stato, la possibilità che qualcuno possa anche sbagliare facendo le cose in proprio e che la certificazione del valore di qualcosa, un titolo di studio, un'impresa, un lavoro, possa venire anche da un giudizio pubblico di una libera società, piuttosto che garantito da uno Stato, che non ha, secondo voi, semplicemente il compito di garantire il rispetto delle leggi per disciplinare il necessario, ma che ha la ben più grave incombenza di stabilire oggettivamente il giusto e l'ingiusto: lo Stato sopra a tutti, quindi lo Stato sopra l'idea, qualsiasi idea di scuola. Siamo così lontani dall'autonomia scolastica, dalla vera libertà, quando si vuole disciplinare ogni cosa. Quindi, per la nostra contrarietà di fondo a questo disegno di legge, come Gruppo dell'UDC, già in Commissione abbiamo avanzato alcune proposte costruttive insieme all'amico Buttiglione. Abbiamo proposto di fermarci, di cominciare un esame serio, uno studio finalizzato all'effettivo funzionamento di tutti i livelli scolastici, di interrompere questa nefasta tradizione la quale vuole che in ogni legislatura una nuova maggioranza provveda a disciplinare di nuovo lo svolgimento dell'esame di maturità. Avevamo proposto di razionalizzare la legislazione vigente e di intervenire, caso per caso, con provvedimenti contenuti e mirati. Proprio dalla relazione a questo disegno di legge abbiamo avuto la conferma di un atteggiamento ben diverso da quello che stiamo auspicando. Si è affermato: «Noi non faremo la riforma di sistema». Bene, ne siamo compiaciuti; non ricominceremo da capo, e questo lo ha affermato anche il ministro Fioroni quando è venuto in audizione nella 7ª Commissione. Ma poi si afferma ancora: «Smonteremo ciò che va smontato, raddrizzeremo ciò che va raddrizzato e adegueremo ciò che va adeguato», e tutto questo naturalmente perché deve essere realizzato «il vero cambiamento utile alla scuola, agli studenti, alle famiglie». È come affermavo prima: non siamo qui appena a fare leggi, cercando faticosamente insieme la strada per ottenere il provvedimento migliore, sentiti tutti, facendoci venire qualche ragionevole dubbio. No, niente di tutto questo, ma una nuova sicurezza, anzi la certezza di una missione quasi evangelica di affermare una nuova verità da parte di una maggioranza che va in piazza contro se stessa, e che vede la manifestazione clamorosa del dissenso all'interno dello stesso Consiglio dei ministri, con voti contrari formalmente espressi. Come fa ad essere così sicura di smontare e raddrizzare e adeguare una maggioranza con così tante divisioni, i cui esponenti sono costretti, in ogni momento, ad invocare il rispetto di quel vangelo laico dell'alleanza di centro‑sinistra, che è il confuso e fumoso programma di Governo? L'un contro l'altro armati nel denunciare il mancato rispetto del documento da cui ogni verità dovrebbe discendere: si faccia ciò che è scritto, secondo la migliore tradizione di ogni società arcaica. Non voglio mettere in discussione la legittimità della maggioranza a governare, fare proposte e cercare di approvarle, ma forse una maggiore umiltà non guasterebbe. Questo linguaggio messianico somiglia molto di più a uno stile *teocon* che a quello *teodem* o *teopop*, al quale facevamo riferimento questa mattina. Se questo è lo spirito con il quale intendete affrontare le cose, non potremo che dare battaglia in modo duro e fermo; se ci sarà un atteggiamento veramente dialogante (come non avete dimostrato in questa occasione), sapremo certamente essere all'altezza di quel contesto più positivo e costruttivo. L'inizio, per quanto riguarda l'istruzione pubblica, non è stata incoraggiante. Non possiamo essere d'accordo con questo disegno di legge, perché volete applicarlo in corso d'anno. Anche questa decisione è frutto di un atteggiamento deterministico e per nulla conciliante. Riteniamo grave questa decisione, perché aumenta lo stato di incertezza nelle nostre scuole. È vero che qualcuno poteva anche sapere, ma non è questa una motivazione seria che si possa presentare in un'Assemblea parlamentare a difesa di questa vostra scelta. Questa decisione non arriverà all'inizio dell'anno scolastico, bensì nel mezzo dell'anno scolastico, a tempo massimo scaduto, per proporre una riforma che comunque cambia in modo sostanziale le regole in campo. Non si cambiano le regole con la partita in corso: questo era il vostro grido di dolore quando il centro‑destra proponeva e approvava la riforma elettorale nello scorcio della precedente legislatura. Questa affermazione non aveva alcun senso in occasione della riforma elettorale, perché non era in corso proprio un bel niente; solo la legislatura era in corso e, finché questa dura, si può approvare qualsiasi legge. Vi abbiamo chiesto di non approvare questa legge; ora vi chiediamo un minimo di buonsenso per non portare in applicazione la legge durante l'anno scolastico 2006-2007: questo sì è veramente in corso. In conclusione, la stessa relatrice ci ha ricordato che negli ultimi undici ci ha ricordato che negli ultimi undici anni, che hanno toccato l'arco di tre legislature, si è provveduto per altrettante volte - tre, appunto - alla modifica della disciplina degli esami di maturità: è veramente troppo, questa ulteriore riforma ce la potevamo proprio risparmiare. Credo, inoltre, che la maggioranza non abbia ben valutato l'impatto di questa normativa. Penso che dovremmo registrare qualche reazione da parte di studenti, famiglie e scuole paritarie avverso questo provvedimento legislativo. Chissà, forse troveremo anche qualche esponente della maggioranza a sfilare contro. Se questo provvedimento verrà modificato in futuro, così da essere reso più ragionevole e più largamente condivisibile, allora potrebbe avere migliori fortune.

Signor Presidente, signora Vice ministro, colleghi e colleghe, nell'annunciare il voto favorevole di Rifondazione Comunista-Sinistra Europea al disegno di legge n. 960, non posso però che partire da una constatazione un po' amara e, cioè, dal fatto che una questione di questa rilevanza è stata seguita con particolare distrazione, non solo da quest'Aula (che, del resto, segue con molta distrazione quasi tutti gli argomenti), ma anche dalla più generale opinione pubblica. In particolare, il sistema dell'informazione ha completamente ignorato questo provvedimento e continuerà ad ignorarlo anche nel giorno in cui esso - come penso - verrà approvato. Da che cosa nasce questa situazione? Penso ci sia una riflessione specifica da portare avanti sui problemi della scuola, che poi sono anche molto concreti, perchè riguardano la vita concreta di milioni di giovani, di famiglie e dell'intera comunità nazionale. Ma la scuola è considerata interessante soltanto se nella misura in cui assume la forma dello scandalo, della cronaca. Un esempio chiarissimo lo abbiamo avuto sotto gli occhi proprio in questi giorni giorni perché tutti gli organi di informazione, i dibattiti televisivi, si sono concentrati su una vicenda alquanto boccaccesca e divertente, anche dal punto di vista concreto. Tuttavia,

che ha strane pratiche sessuali con i suoi allievi, è stata considerata, perfino in quest'Aula, dal senatore Asciutti, come una vicenda in qualche modo esemplare, significativa, o comunque rappresentativa dello stato della scuola italiana quando è invece evidente che siamo di fronte ad un episodio circoscritto. Oppure, per fare solo un altro esempio, la scuola fa notizia e diventa un tema interessante se qualcuno, come si usa fare con una certa frequenza in questa fase, spiega che gli insegnanti sono sostanzialmente una massa di lavoratori nullafacenti e privilegiati e se un'esponente

Potrei continuare a lungo, ma ovviamente andrei fuori tema. Vorrei solo utilizzare questa occasione, che pure è stata importante, per ricordare a tutti noi che stiamo parlando di questioni che hanno a che fare

rivolgo al senatore che mi ha preceduto: se una legge viene fatta e rifatta molte volte significa che c'è in essa qualcosa che non funziona e, comunque, non si tratta di una valida ragione per lasciare le cose come stanno. Corregge il sistema dell'istruzione in un punto chiave che è quello di restituire valore all'esame di Stato e al titolo di studio.

una tendenza qualunque e innocente; è parte integrante e una delle conseguenze meno innocenti della pratica neoliberista che tende a deprimere

mobilità sociale che ha caratterizzato l'Italia nell'ultimo scorcio di quello che il grande storico Hobsbawn ha chiamato «Il secolo breve», quando le masse popolari sono riuscite a entrare nella scuola e il sistema dell'istruzione ha assunto una diversa portata e un diverso valore.

La questione della legge di parità è tornata in questo dibattito. Voglio solo farvi un accenno: noi non l'abbiamo condivisa allora e continuiamo a nutrire delle riserve.

che ci è caro e spinge a considerare il primato dell'istruzione pubblica sulla privata. È qualche cosa di più significativo

È un fatto su cui forse, anche all'interno della coalizione di maggioranza di cui facciamo parte, sarà bene sviluppare una riflessione approfondita per fare un bilancio della suddetta legge a sei anni dal suo funzionamento.

non può essere soggetta a una logica merceologica. La conoscenza ha senso, si arricchisce, assume anche una funzione di promozione democratica soltanto e nella misura in cui diventa un elemento di diffusione

qual è la differenza tra la destra e la sinistra, tra il Governo precedente e quello attuale anche sugli esami di maturità? noi, anche con le nostre differenze e le nostre articolazioni, pensiamo ad una scuola per tutti, a una scuola di qualità per tutti. Chi pensa ad un'idea di scuola elitaria o per le classi dirigenti, come è stato fino ad una lunga fase della storia umana, fa presto a fare una buona scuola o una scuola eccellente. Fare una buona scuola una buona scuola alla quale tutti e tutte possano accedere è per noi non solo un grande problema di strategia politica e culturale, ma è uno dei cardini della nostra democrazia. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che anche la maggioranza possa dare atto ad Alleanza Nazionale di aver svolto un'opposizione costruttiva. Noi abbiamo scelto deliberatamente di non ricorrere a forme ostruzionistiche, perché riteniamo che la scuola sia un bene comune che non può essere oggetto di una battaglia politica di parte. Ciò ovviamente non toglie che

questo è il senso della riforma Moratti e dell'atteggiamento di Alleanza Nazionale in questo dibattito che è stato certamente, e soprattutto in Commissione, anche molto alto.

sei studenti su dieci non sono riusciti a calcolare l'aumento percentuale di due bollette della luce. Vi ho letto ieri risultati particolarmente inquietanti, secondo

La scuola che esce da questa riforma è sempre la solita scuola: è mancato un colpo d'ala. Ci saremmo aspettati ben altro, ci saremmo aspettati delle vere novità.

Parliamoci chiaro: la nuova disciplina sugli ottisti, cioè i ragazzi che saltano l'ultimo anno, le norme di contrasto ai cosiddetti diplomifici, la reintroduzione dello scrutinio di ammissione alla maturità, il fatto che i debiti formativi debbano essere scontati per potere accedere alla maturità, il rapporto con il mondo dell'università, sicuramente molto più organico nella legge Moratti, la legge n. 53 del 2003, tutto questo lo avevamo già approvato noi. Cari amici, Cari amici, alcuni di voi non c'erano nella passata legislatura. Sappiate che in Commissione si è discusso molto, ma erano misure già contenute nel decreto Moratti che - ripeto - voi avete sospeso.

a quella norma che prevede che i commissari esterni siano sostanzialmente della stessa area. Stamattina vi ho letto il testo dell'ordine del giorno firmato da me e dal senatore Ranieri

regionali. In definitiva, ci aspettavamo una riforma che non fosse precaria, transitoria. Dal dibattito in Commissione, ma anche da alcune dichiarazioni espresse dal vice ministro Bastico, emerge invece che questa riforma dovrà essere in qualche modo ritoccata, quando si affronterà il problema della riforma delle superiori.

un tentativo di compromesso per venire incontro alle esigenze dell'opposizione e a quelle della maggioranza, che invece andavano in senso diverso (tranne forse qualche persona più illuminata). più illuminata). Dobbiamo volere una scuola che responsabilizzi veramente. Per esempio, mi ha stupito che in Commissione si sia tentato di lanciare il sasso, e nessuno abbia approfittato di quegli emendamenti dell'opposizione che stabilivano un limite di assenze per accedere alla maturità, per affrontare un problema che in Italia viene sempre messo sotto il tappeto. Siamo l'unico Paese al mondo ad avere le occupazioni delle scuole come dato permanente nel nostro sistema scolastico: la scuola *happening*. Credo non se ne possa più.

di affrontare questo problema, perché problema di serietà della scuola. Allora, perché non approfondire? Perché non prendere spunto da qualche elemento positivo che pure traspare ogni tanto nel mondo culturale che vi accompagna? Senatore Ranieri, lei è persona troppo intelligente per non capire che le vostre divergenze sono molto diverse da quelle differenze di posizioni che si sono manifestate nel dibattito, per esempio, tra noi e Forza Italia. Forza Italia ha preferito la scelta dei commissari tutti interni per rivendicare una continuità che, peraltro, era frutto di un mero calcolo contabile, esattamente come voi non avete avuto il coraggio di scegliere i commissari tutti esterni, perché certamente costano, perché sono riforme costose. Ma quando voi scegliete di dire no alla valutazione o di discriminare

concludere, dobbiamo guardare seriamente al futuro. Ma cosa possiamo fare insieme per la scuola italiana? Quando dissi che Alleanza Nazionale era disponibile a ragionare,

di stipendi finalmente legati al merito? Perché tutti gli insegnanti devono essere pagati allo stesso modo, sia che lavorino seriamente e si autoaggiornino sia che non facciano nulla? Perché non varare un serio sistema di valutazione delle scuole? Perché non varare un'area contrattuale separata, come la parte avanzata del sindacato rivendica, per distinguere e nobilitare gli insegnanti rispetto al personale, per esempio, non docente, che svolge un ruolo fondamentale, ma che deve avere deve avere altre situazioni contrattuali dal punto di vista della base di riconoscimento giuridico? Perché non incoraggiare l'autoaggiornamento? Perché non andare verso quel *budget* di istituto che è una grande conquista di molti altri Paesi occidentali? Questi sono problemi seri. Temo però che, nonostante qualcuno di voi sia disponibile a confrontarsi, queste proposte rimarranno sul tavolo, perché da parte vostra, purtroppo, non c'è una maggioranza culturalmente in grado di affrontare seriamente i problemi della scuola italiana.

In premessa vorrei ricordare quel che è accaduto con il decreto Bersani-Visco, o meglio, Visco-Bersani. Si è parlato per un mese intero dei tassisti, poi, alla fine, abbiamo scoperto le nefandezze della legge Visco, che a suo tempo fu detta Bersani.

in base alle loro possibilità (e quindi sono aperte tutte le varie possibilità, nel senso che da un istituto possono passare ad un altro e l'obbligatorietà può essere anche effettuata nella formazione professionale), oppure

è fuor di dubbio che, in sede di Commissione, tanti emendamenti dell'opposizione, compresi i miei e quelli del mio Gruppo, sono stati accettati dalla maggioranza; ma vi ricordo che non è un favore che avete fatto voi a noi,

di politica seria, non sono stati accettati né in Commissione, né in quest'Aula. Veniamo ad un altro punto. Mi ricordo che

Ditemi di una riunione che avete fatto con qualcuno. Avete parlato forse con i ragazzi che ci stanno ascoltando dalle tribune qui sopra? No. Avete parlato con qualche istituzione scolastica? No. Avete convocato qualcuno? No. Questa è la realtà:

in campagna elettorale di bugie se ne dicono tante, e voi sapete come si dicono. Il problema - ripeto - non è l'esame di Stato. Il problema è ormai storico per questo Paese: bisogna invertire la tendenza negativa delle nostre scuole. La tendenza negativa delle nostre scuole è che c'è poca serietà negli studi, poca serietà negli apprendimenti, poca serietà nel contesto sociale nei confronti della scuola. che oggi la scuola è quasi un parcheggio; che lo studente studi o meno, non cambia nulla. Il problema è che non bisogna disperdere nessuno, come all'università. Per non disperdere nessuno e far sì che le statistiche si alzino, dobbiamo promuovere tutti. non facciamo assolutamente il bene né degli studenti, né della società, né di questo Paese.

mi rimproverava di aver preso come spunto un fatto, che spero anch'io essere un fatto unico. Ma il problema è un altro: non c'è più, nella società, quel senso di sacralità nei confronti della scuola che un tempo c'era. È lì il problema: l'abbiamo completamente distrutto. Allora bisogna tornare ai valori di un tempo. *(Applausi dal Gruppo* *FI)*. Oggi, purtroppo, nella scuola si dice che è tutto permesso, è tutto consentito, in nome di una falsa libertà.

Altri due punti e finisco, signor Presidente; si è tornati in quest'Aula, come in Commissione, ad accentuare quello sterile pregiudizio tipico di una certa sinistra nei confronti delle scuole paritarie. avviso, per gli studenti deve essere libero l'accesso al servizio pubblico di istruzione e, quindi, sia alle scuole statali che a quelle paritarie, senza distinzione e senza pregiudizi. La La senatrice Pellegatta ricordava la legge di parità; no, lei può essere contro la legge di parità e comprendo, come dice la Gagliardi, ma la legge di parità è chiara. pone allo stesso livello, come l'articolo 33, terzo comma, della Costituzione prevede, sia le scuole paritarie che le scuole non statali che fanno entrambe parte, senatrice Gagliardi, del servizio pubblico di istruzione. Non confondiamo statale con pubblico perché anche le scuole paritarie fanno parte del servizio pubblico. Il problema, poi, significativo e culturale che era fondante di una riforma dell'esame di Stato, che metteva in discussione negli anni precedenti il tutto, era la famosa terza prova che anche voi avete compreso, accettando in parte l'emendamento dell'opposizione, ma non accettandolo nel suo complesso. Se non andiamo avanti con la terza prova per mettere in condizioni di comprendere che ciò che è fondamentale sono le conoscenze dei saperi e non il nozionismo, non riusciremo a modificare il livello culturale del Paese; è questa la realtà delle cose. Avete appena accolto, quasi come fosse un ordine del giorno o poco più, in legge, questo nostro pensiero; ma non è un nostro pensiero, è il pensiero dell'Europa. Noi siamo fuori dell'Europa. Come del resto siamo fuori dell'Europa - non me ne vogliate - per l'obbligatorietà del valore legale del titolo di studio. Siamo, forse con l'Argentina, gli unici Paesi al mondo che hanno il valore legale del titolo di studio. Non è un problema, perché che ci facciamo con il valore legale del titolo di studio? Dovete spiegarmi che cosa ci facciamo! Almeno, a quel punto, riesco a capire il significato forte del valore legale del titolo di studio, oggi, in questo Paese.

dove nulla è consentito all'opposizione di ottenere perché altrimenti il popolo, gli elettori, non capirebbero.

Giustamente, qualcuno mi suggerisce di ricordare che gli elettori sono seri e non sono assolutamente pazzi, come il vostro capo del Governo va tutti i giorni dicendo. *(Applausi del

Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo svolto una discussione intensa e seria sulla scuola che finalmente è entrata in quest'Aula e ha visto riconosciuta, in questi giorni di dibattiti, la dignità e l'importanza che ha nella società del nostro Paese. Abbiamo presentato una riforma che aveva l'obiettivo fondamentale di restituire serietà all'esame di maturità, di rispondere ad un allarme rispetto all'esame di maturità che era stato provocato da un'improvvida riforma del Governo di centro-destra, quello che rendeva che rendeva tutti interni i membri delle commissioni. Una riforma che ha provocato abusi pesanti. Io vedo solo una cifra,

lo 0,4 della popolazione di riferimento. Dopo la riforma Moratti sono diventati 19.040, il 26,9 della platea di riferimento.

maturità. Rispetto a questa situazione si erano indignate non solo le scuole pubbliche ma anche le scuole paritarie serie. Leggete il documento della Federazione italiana delle

perché abbiamo condiviso in Commissione, come anche con voi, un percorso di costruzione unitaria del disegno di legge. E' il disegno di legge di tutta la maggioranza, e per alcuni aspetti ha ricevuto anche un vostro contributo importante e significativo.

superiore. I Paesi più seri sono quelli con i più alti livelli di apprendimento e il più basso livello di dispersione. In Finlandia, i cui risultati OCSE citate sempre per dimostrare quanto brutta sia la scuola italiana, ha alti livelli di apprendimento ma diploma il 93 per cento degli iscritti in prima superiore: questa è la serietà che bisogna acquisire. Una scuola inclusiva è una scuola seria. È questo l'obiettivo cui tendere,

La scuola italiana è messa sotto accusa dall'OCSE-PISA perché non solo abbassa i rendimenti medi, ma anche perché ha il più basso indice di equità. E' un sistema scolastico in cui le differenze non dipendono dalle differenze tra gli individui, ma dal tipo di scuola cui si è iscritti. Le eccellenze sono tutte per il liceo, mentre i punti bassi sono tutti per l'istruzione e la formazione professionale. A questo bisogna porre rimedio e costruire un'idea del merito che, eviti di essere contrassegnato da divisioni classiste. Per questo siamo per il biennio unitario, che non vuol dire unico, ma che mette insieme il sapere e il saper fare; che integra i saperi, ma che punta a non rendere irreversibile e rigida la scelta, che poi si riproduce puntualmente nei livelli di apprendimento dei ragazzi a seconda della scuola frequentata. Di questi argomenti ha finalmente cominciato a parlare Draghi, non i pedagogisti: l'altro giorno, intervenendo al convegno Unioncamere, ha detto che la scuola è il tallone d'Achille della competitività del Paese e che intervenire sulla scuola è assolutamente necessario; su quella scuola che voi avete governato per cinque anni e noi per cinque anni prima. Basta darsi le colpe! Diciamo che bisogna intervenire, senza citare i risultati dell'OCSE-PISA come fosse colpa di Berlinguer. Credo che dopo sei mesi si debba smettere di dare la colpa al Governo precedente.

il decreto Bersani, tentativo, quest'ultimo, di spostare in avanti la qualità delle imprese e la capacità delle imprese di internalizzare il sapere, di abbattere le barriere corporative al merito che esistono nel sistema delle professioni.

Colleghi, la seduta non è sospesa, è ancora in corso.

Grazie,

rivela che l'esame del progetto di legge comunitaria risenta di varie strette. La stretta temporale, innanzitutto. Il cambio di legislatura e la pausa elettorale hanno fatto sì che questa legge sia figlia di due differenti Governi e giunga con grave ritardo all'appuntamento annuale. la stretta determinata dal peso di un contenzioso comunitario sempre oscillante, purtroppo, ad un livello inaccettabile per un Paese che ha mantenuto un indirizzo politico costantemente orientato, almeno sul piano normativo, ad una piena adesione agli obiettivi comunitari. Se guardiamo, infatti, alle procedure di infrazione, 102 sono le messe in mora, 73 i pareri motivati e 42 i ricorsi già avviati alla Corte di giustizia;

la stretta che possiamo definire storica, determinata dal mancato adeguamento dei Regolamenti della Camera e del Senato a quel modello di procedura sagomato sulla legge finanziaria che da anni pur si ripete di voler perseguire, sia per quanto riguarda i vincoli propri di sessione, sia per quanto riguarda l'unificazione di fasi conoscitive tra Camera e Senato. In sostanza, signor Presidente, con la legge comunitaria abbiamo inventato uno strumento giuridico pressoché unico negli ordinamenti nazionali dell'Unione Europea, ma non gli abbiamo fino ad ora dato un adeguato e completo seguito regolamentare e parlamentare, alla fine dei conti, risultano più efficaci ordinamenti che non hanno procedure complessive come quella della legge comunitaria, ma dispongono nel loro ordinamento costituzionale di un'automatica delega implicita per l'attuazione delle direttive comunitarie. Tutte queste strette temporali e procedurali, temperate peraltro dall'assicurazione del Governo di voler al più presto presentare in Parlamento un primo schema della prossima legge comunitaria, hanno fatto sì che la Commissione referente si sia posta un autolimite nella ricezione di emendamenti, anche rispetto ad emendamenti utili in linea di principio ed ammissibili. Questo lavoro si è innestato, signor Presidente, su un progetto di legge comunitaria con cui la Camera dei deputati ha apportato decisive innovazioni nella serie di obblighi di informazione da parte del Governo al Parlamento, che riguardano le procedure di contenzioso e di precontenzioso in relazione alle sentenze della Corte di giustizia e le procedure di infrazione ed obblighi di informazione che riguardano anche l'andamento dei flussi finanziari tra l'Italia e l'Unione Europea, andamento che sarà oggetto di una relazione trimestrale al Parlamento. È quindi un adeguamento informativo pieno, con spunti addirittura di avanguardia, del nostro sistema parlamentare a quel movimento assai diffuso che tende ad avvicinare sempre più i Parlamenti nazionali alle procedure decisionali dell'Unione. Anche per queste ragioni di politica istituzionale e comunitaria le nostre considerazioni iniziali sulla migliore collocazione istituzionale della legge comunitaria nell'economia dei lavori parlamentari meritano un'attenzione assai più viva che nel passato. organizzazione del nostro lavoro sulle scelte di politica europea, ormai così invasive in ogni angolo delle nostre procedure, meriterebbe migliore collocazione anche la relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea che la collega Soliani

che mi accingo ad esporvi in modo sintetico, illustra l'attività svolta dal Governo nelle varie politiche dell'Unione nel 2005 e indica gli orientamenti per il 2006.

registriamo i passi che abbiamo fatto e che stiamo facendo ed anche i problemi aperti. Faccio notare che la Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'attività dell'Unione nel 2005, con gli orientamenti per il 2006, giunge all'esame del Parlamento con notevole distanza dalla sua elaborazione; pertanto, in alcune parti essa non risulta aggiornata. Tuttavia, vorrei far notare il dato politico. La Relazione attraversa il crinale tra due legislature, con Governi di segno politico diverso e l'*iter* ha risentito delle elezioni per il rinnovo delle Camere. È naturale che si possano registrare anche approcci differenti, ma in ogni caso il Ministro per le politiche europee sta già provvedendo, nelle competenti sedi, ad illustrare i punti qualificanti del programma e dell'azione dell'attuale Governo in ambito europeo. Tuttavia, questa è l'occasione per ribadire, in questo passaggio politico e democratico, che la consapevolezza delle attuali difficoltà dell'Europa richiede l'impegno comune di tutto il Parlamento, oltre che del Governo, per rilanciare il processo di costruzione politica e costituzionale dell'Europa, nel solco della storia politica del nostro Paese, cinquant'anni dopo i Trattati di Roma. Siamo qui per ricordare, con un'assunzione di responsabilità che abbraccia questo arco temporale e maggioranze diverse, che l'iniziativa dell'Italia e più che mai necessaria. Nella relazione si toccano i punti essenziali attorno a cui si è mossa l'azione politica del Governo e del nostro Paese. Innanzitutto, il processo di integrazione europea e la riforma costituzionale, che ha subito una battuta d'arresto con l'esito negativo dei *referendum* in Francia e in Olanda. Il Governo italiano ha sostenuto la decisione del Consiglio europeo di avviare un periodo di riflessione sul Trattato costituzionale. Ci aspettiamo, in vista delle elezioni del 2009 per il Parlamento europeo, di poter arrivare a un completamento della riforma costituzionale. Pensiamo che anche le celebrazioni del prossimo 25 marzo 2007 a Berlino e a Roma, nell'anniversario della firma dei Trattati, possano essere l'occasione per una ripresa molto forte della volontà politica degli europei di giungere alla riforma costituzionale per rafforzare il processo di integrazione. Altro tema strategico è quello dell'allargamento. L'Italia ha sostenuto l'adesione della Romania e della Bulgaria, che entreranno nell'Unione Europea il 1° gennaio 2007, nonché l'avvio dei negoziati con la Turchia e la Croazia.

ma abbiamo anche potuto registrare la loro grande riconoscenza verso l'Italia, che ha sempre sostenuto la loro adesione. Sulla relazione abbiamo raccolto i pareri delle diverse Commissioni del Senato e dobbiamo sottolineare che anche da esse è venuta la spinta per ulteriori riflessioni ed impegni.

così come sosteniamo fermamente la necessità di una politica estera efficace, perché, evidentemente, nel mondo c'è bisogno dell'Italia, ma c'è molto bisogno di Europa. terzo tema strategico concerne la Strategia di Lisbona, una sorta di bussola dell'ultimo decennio. Dobbiamo dire onestamente che l'Europa non ha fatto tutti i progressi che si sperava sulla Strategia di Lisbona in quanto siamo già oltre la metà del decennio, con gli obiettivi posti al 2010. Tuttavia, dobbiamo registrare - la relazione lo registra - il Piano per l'innovazione, la crescita e l'occupazione, denominato PICO (il riferimento è, ovviamente, al grande Pico della Mirandola,

Su questo debbo dire che il ministro Bonino è stata molto tempestiva e, pur avendo assunto l'incarico pochi mesi fa, ha tenuto fede alla data che prevedeva il rapporto dell'Italia sul Piano PICO. Alti temi importanti sono l'innovazione tecnologica, il versante della ricerca in tutti i comparti industriali e una speciale attenzione al settore energetico. In questo senso si è espressa la Commissione industria. Sul tema della formazione e del lavoro, siamo invitati ad una particolare attenzione al tema della formazione e della valorizzazione del capitale umano, coerentemente con gli orientamenti dell'Unione Europea. Grande attenzione, ancora, in ragione dei cambiamenti demografici, va posta ad interventi finalizzati alla creazione di posti di lavoro più numerosi e più qualificati, naturalmente favorendo la promozione di politiche di contrasto alla disoccupazione di lungo periodo e giovanile e l'attuazione di misure per la regolarizzazione del mercato del lavoro e dei sistemi pensionistici. Possiamo dire che tutta la realtà dei temi più forti e più problematici della nostra società (che è italiana e insieme europea) è davvero affrontata.

la proposta di regolamento per istituire un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, mirato al reinserimento professionale dei lavoratori in seguito a importanti modifiche strutturali nel commercio mondiale. poi una forte attenzione alle nostre politiche nel settore della libertà, sicurezza e giustizia, perché dobbiamo dare attuazione al cosiddetto programma dell'Aja. occorre prestare attenzione alla proposta di revisione della direttiva sulla cosiddetta TV senza frontiere. Come vedete, vi sono altri temi che per brevità non tocco, ma la relazione traccia un quadro molto attuale ed esaustivo dei principali problemi di fronte ai quali si trova il nostro Paese in relazione alle politiche dell'Unione Europea. La relazione, infine, dà conto della situazione riguardante le procedure di infrazione (sappiamo che questo è un terreno per noi assai problematico),

e quelle (in numero invece più elevato) dovute a violazioni del diritto comunitario. Abbiamo la necessità di migliorare l'adeguamento delle norme nazionali al diritto comunitario. Abbiamo bisogno che ci sia un'importante partecipazione dell'Italia all'adeguamento amministrativo con la cultura europea, perché dobbiamo velocemente, anche in termini culturali, affrontare il tema delle infrazioni. Infine, appare particolarmente apprezzabile la trasmissione da parte del Ministro del commercio internazionale del rapporto della Commissione europea sulle decisioni adottate il 12 ottobre 2006 relative alle infrazioni inerenti all'Italia. all'Italia. Per la seconda volta, dobbiamo dare atto al Ministro della tempestività con la quale rappresenta il nostro Paese nell'Unione Europea, anche quando tale rappresentanza fa toccare i problemi concreti delle nostre inadeguatezze.

Lei sa, signor Presidente, qual è il valore e l'importanza dei grandi dibattiti che sulla politica europea si devono svolgere nei Parlamenti perché insieme col Parlamento europeo anche questi abbiano un ruolo di indirizzo e di guida del Governo.

Se fossi in vena di fare della retorica e non fossi moderato, direi che oggi il Parlamento italiano rischia di rendersi colpevole del reato di vilipendio delle istituzioni europee. È un momento in cui la crisi della politica europea sta raggiungendo un livello di massima in cui dovremmo tutti interrogarci sul modo di far ripartire l'ideale europeista. È un momento in cui sono di fronte a noi scelte politiche europee di altissimo rilievo e importanza: dall'ingresso della Turchia - come voi sapete, oggetto di forte dibattito - al modo di far ripartire il processo costituzionale europeo. È un momento in cui gran parte della normativa che effettivamente tocca la vita della gente si produce in Europa. Negli Stati nazionali si distribuiscono i denari, ma le leggi ormai si fanno, per il 33 per cento delle norme di rilievo, a livello europeo. Abbiamo in programma una grande riforma del mercato dei servizi, la cosiddetta direttiva Bolkestein (di cui, peraltro, Bolkestein rifiuta la paternità); c'è una questione di politica industriale, da cui dipende il futuro dell'industria chimica in Europa, come il REACH. di tutto ciò con interventi contingentati di quattro o cinque minuti, in un'Aula che chiaramente, per giuste ragioni, è estenuata e non ha la capacità di concentrare l'energia nervosa necessaria per affrontare queste grandi questioni politiche.

Signor Presidente, mi pare che il senatore Selva nel suo intervento abbia di fatto posto una questione sospensiva,

intende considerare il suo intervento sull'ordine dei lavori nel senso di una questione sospensiva, mi pare sia questo il momento per farlo.

Grazie, Signor Presidente, l'ordine del giorno da me presentato è un invito al Governo ad adempiere ad alcuni impegni economici già acquisiti in relazione alle politiche comunitarie in favore della gioventù per il periodo 2007-2013. Coerentemente con il principio di sussidiarietà contemplato dal Trattato di Nizza, molte delle azioni promosse dai programmi comuni*«*LifeLong Learning» e «Gioventù in Azione» prevedono un cofinanziamento dei costi di realizzazione delle attività, demandando allo Stato membro le iniziative necessarie per garantire il regolare funzionamento dei programmi. Considerato che, se non verranno messe a disposizione le risorse logistiche ed economiche volte a dare efficienza ai programmi sopracitati e a garantire l'adeguato cofinanziamento per le specifiche azioni in cui esso si rileva come obbligatorio, non sarà possibile per i giovani e gli operatori partecipare a tali opportunità, questo ordine del giorno impegna il Governo a garantire la piena accessibilità dei giovani e degli operatori ai programmi dell'Unione Europea «Gioventù in azione» e *«*LifeLong Learning», anche al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi posti dalla Strategia di Lisbona, garantendo altresì, attraverso autonomo provvedimento, ovvero nel contesto della formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, la piena disponibilità delle risorse necessarie a cofinanziare i predetti programmi.

al problema dei rifugiati, al titolo di soggiorno da rilasciare a cittadini di Paesi terzi vittime della tratta di esseri

alla direttiva MiFID e alle modifiche intervenute sulla legge sul risparmio. Abbiamo manifestato molte perplessità per la decisione del Governo di utilizzare questo strumento per cancellare alcune norme della legge sul risparmio. Intervengo per illustrare un ordine del giorno che può rappresentare un momento marginale rispetto alla complessità dei temi e che tuttavia pone in rilievo una questione di un certo interesse. Con la legge 23 giugno 2000, n. 178, il Governo italiano è stato autorizzato a stipulare un'intesa con la Commissione europea, al fine di istituire il Centro nazionale di informazione e documentazione europea La Commissione europea, con decisione del 28 novembre 2005, ha ritenuto di non rinnovare la sua partecipazione ai Centri nazionali di informazione sull'Europa per sopravvenuta incompatibilità con le disposizioni del proprio regolamento finanziario. Con la medesima decisione la Commissione, in coerenza con il Piano d'azione del 20 luglio 2005, offre ai Governi dei Paesi membri e, in particolare, alla Repubblica francese, alla Repubblica del Portogallo e alla Repubblica italiana, nuove forme di collaborazione definite «partenariati di gestione», nelle quali è, tra l'altro, previsto di poter eventualmente anche utilizzare lo strumento collaudato dei Grandi Centri per far fronte alle esigenze di informazione dell'opinione pubblica sulle attività dell'Unione Europea in maniera coordinata e permanente. II contratto istitutivo del CIDE prevede che un membro fondatore possa domandare proroga della durata del gruppo europeo di interesse economico. I Governi francese e portoghese hanno richiesto la proroga dei rispettivi contratti per permettere di avere più tempo per trovare nuove fondamenta giuridiche e finanziarie per le loro rispettive strutture. La Commissione europea ha già espresso anche al Governo italiano la sua disponibilità a convenire su una siffatta proroga al fine di procedere alla trasformazione del Centro su nuove basi giuridiche, nonché per migliorarne

Dicevo, per migliorarne ulteriormente l'idoneità quale strumento di informazione e comunicazione europea secondo le modalità indicate dal Piano d'azione SEC(2005)985 e dal Libro bianco su una politica europea di comunicazione.

da un lato di disperdere un *know-how* e una professionalità ormai acquisite, dall'altro significa l'implicita rinuncia da parte del Governo italiano a ripristinare, se non in tempi lunghissimi, un corrispondente strumento d'informazione europea con analoghe responsabilità a livello nazionale. Proprio in un momento in cui tutti gli Stati membri dell'Unione proclamano di voler aumentare gli sforzi per avvicinare i cittadini al processo di integrazione europea. Queste considerazioni rappresentavano un appello al ministro Bonino affinché non si disperda e non si smantelli questa struttura e si consenta di proseguire su un cammino che possa essere utile al Paese.

tutto ciò che aveva già previsto lo stesso disegno di legge del Governo Berlusconi, sia perché trattavasi di atto dovuto sia per evitare ulteriori ritardi nel recepimento di direttive comunitarie.

sono riusciti a ridurre, negli ultimi tre anni, le procedure di infrazione per rimanere al di sotto della soglia del 50 per cento relativa al 2006.

il parere del Governo), per quanto concerne in particolare il controllo delle attività di consulenza delle società di credito, delle banche, delle società finanziarie e delle società di assicurazione. Con un emendamento approvato in Commissione all'unanimità è stata eliminata la norma che, nel testo approvato dalla Camera, cancellava la qualifica professionale privata di circa 7.000

vorrei ricordare che il testo in esame, che noi stiamo per approvare, non ripropone due previsioni contenute nelle ultime leggi comunitarie, con cui si introduceva la trasmissione, da parte del Ministro per le politiche europee, di una relazione al Parlamento, qualora una o più deleghe conferite dalla legge comunitaria non risultasse esercitata trascorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione, nonché di un'informativa periodica quadrimestrale sullo stato di attuazione da parte delle Regioni e delle Province autonome. Il comma 6 dell'articolo 1, signor Ministro, che reca invece una significativa novità rispetto ai contenuti consueti, autorizza il Governo, entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi adottati per il recepimento di direttive per le quali la Commissione europea si sia riservata di adottare norme di attuazione, a recepire tali disposizioni allorché effettivamente adottate con regolamenti governativi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988. Così come pure il comma 7 dell'articolo 1 richiama l'applicazione della consueta clausola di cedevolezza,

citata legge n. 11 del 2005. Pertanto, le precedenti leggi comunitarie recano una disposizione che prevedeva un intervento suppletivo anticipato e cedevole, da parte dello Stato, in caso di inadempimento delle Regioni e in caso di attuazione dei provvedimenti stessi. Queste sono le norme sostanziali più evidenti a cui facciamo riferimento in questo provvedimento, che naturalmente richiama centinaia di norme, e credo che il Governo,

che prevedeva la presenza di traccianti colorati nel latte in polvere destinato ad uso zootecnico perché questo non potesse essere confuso con latte ad uso umano. Oggi la norma comunitaria ci chiede di abrogare questa legge e quindi di evitare, come si era previsto, che dei prodotti caseari, come il latte, vengano arricchiti con il latte in polvere ad uso zootecnico o che - come troppe volte purtroppo è successo - questi tipi di latte ad uso zootecnico possano essere commerciati nei Paesi impoveriti,

Signor Presidente, signor Ministro, gentili colleghi, il disegno di legge che ci accingiamo a votare è parte fondamentale ed essenziale della vita del Paese. Non si tratta di mero rituale,

Il nostro Paese riceve dall'Unione Europea una parte consistente della sua legislazione, che concorre però a formare in sede comunitaria. Questo processo è di tipo federale, ma oggi ancora incompleto e insoddisfacente. Questa incompletezza e l'accusa, non sempre infondata, di opacità nel processo decisionale permettono e talvolta invitano ad attacchi contro il*deficit* democratico di cui patirebbe l'Unione Europea e contro l'eccessiva burocratizzazione della Commissione europea. Occorre quanto prima porre rimedio a questa situazione agendo su due fronti: la ripresa del processo di integrazione europea e una maggiore attenzione alla trasparenza degli atti comunitari. La riforma e il rilancio del processo di costruzione europea sono già tra le priorità del Governo, e siamo fiduciosi che questo saprà infondere nuova e determinante energia e convinzione, insieme con Francia e Germania che si divideranno la Presidenza di turno dell'Unione Europea nel 2007, anno in cui ricorrerà il cinquantesimo anniversario della firma del Trattato di Roma. Spero, l'anno prossimo, di poter votare su una legge comunitaria che porti già in sé le tracce di un nuovo inizio dell'azione dell'Unione Europea. Maggiore trasparenza e maggiore senso di responsabilità sono invece possibili anche a livello di singoli Stati membri. E mi parrebbe giusto che l'Italia desse in questo senso un buon esempio.

Il vantaggio di disporre di tempi sicuri per l'approvazione della legge comunitaria e della relazione annuale avrebbe il grande merito di accordare, anche formalmente, il giusto peso ad atti fondamentali per la vita del Paese. Il dibattito che ne scaturirebbe sarebbe l'occasione per le forze politiche di illustrare apertamente alla popolazione le proprie posizioni su temi di altissimo impatto sulla loro vita. Non dimentichiamo che una direttiva comunitaria spesso può cambiare la vita degli italiani molto più di un emendamento alla legge finanziaria sulla quale, come è noto, il dibattito e le prese di posizione sono accesi ed oltremodo pubblicizzati. Nel merito di questa legge comunitaria sottolineo, anche alla luce di quanto detto, alcuni aspetti che giudichiamo estremamente positivi. Innanzitutto, l'introduzione intervenuta alla Camera di un Capo II che prevede obblighi di informazione da parte del Governo al Parlamento sulle procedure di contenzioso e precontenzioso nei rapporti con l'ordinamento comunitario, sulle sentenze prodotte dalla Corte di giustizia, sulle procedure di infrazione nonché sull'andamento dei flussi finanziari tra l'Italia e l'Unione Europea. Trattasi, giustamente, di un passo significativo ed apprezzato nella direzione di una maggiore trasparenza, pur con le modifiche subite. Fondamentale è l'aggiunta del Capo III, recante i princìpi fondamentali nel rispetto dei quali le Regioni dovranno esercitare la propria competenza normativa e relativi alle materie della legislazione concorrente attinente alle direttive contenute negli allegati al disegno di legge. Nuovamente, si tratta di una misura volta a fare chiarezza e ad evitare inutili contenziosi ma, soprattutto, è il riconoscimento formale del ruolo fondamentale delle Regioni nell'architettura della costruzione europea. più destinatarie in seconda battuta di una legislazione europea, che apparirebbe così sempre più distante, ma soggetti attivi e cooperativi con i livelli nazionale ed europeo. Provengo da una regione di confine e posso testimoniare quanto queste realtà plurilingui, collegamento tra culture diverse piuttosto che limiti invalicabili come nel passato, abbiano ritrovato un ruolo e una feconda libertà nella costruzione di un'Europa unita. Annuncio, pertanto, il voto favorevole del Gruppo per le Autonomie oltre che il mio, rinnovando una volta l'augurio che l'Italia riprenda il percorso di una costruzione europea convinta e, perché no, entusiasta.

G103 impegna il Governo innanzitutto all'attuazione degli articoli 5 e 6 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'agricoltura e l'alimentazione. Se la signora Ministro potesse prestarmi ascolto, vorrei dire che con rammarico

e l'alimentazione, la questione a livello italiano e internazionale ha molto a che fare con i problemi della fame nel mondo e la conservazione è l'oggetto Purtroppo, le tendenze del mercato delle sementi fanno sì che si vada sempre di più verso la standardizzazione con gran parte di cloni, che hanno ovviamente ridottissime variazioni. legislazione non prevede ancora, purtroppo, la possibilità del recupero e del mantenimento delle varietà a rischio. Solo i semi iscritti al catalogo ufficiale possono essere commercializzati. Inoltre, la nostra disciplina vieta ancora l'utilizzo e lo scambio tra agricoltori di sementi non registrate. Questo ha fatto sì che

agli articoli 5e 6 del Trattato, che prevedono appunto la necessità, per i Paesi che lo hanno sottoscritto, di misure volte a tutelare lo scambio delle sementi e la biodiversità. Faccio anche riferimento al bellissimo manifesto

a questi impegni: provvedere all'istituzione di un apposito registro nazionale nel quale siano iscritte le varietà a rischio di erosione genetica; che l'iscrizione sul suddetto registro sia gratuita ed esentata dall'obbligo di esame; riconoscere ai produttori agricoli, residenti nei luoghi dove le varietà di cui sopra hanno evoluto le loro proprietà

Una lamentela ricorrente che riguarda il nostro Paese è che siamo il fanalino di coda nel processo di attuazione della normativa comunitaria. Spero di essere smentito, ma mi pare che oggi siamo il venticinquesimo Paese su 25 giù di lì. si consenta di ricordare che non è sempre stato così. Tra il 2001 e il 2004, per esempio, l'Italia - che era il quindicesimo di 15 Paesi, è risalito fino ad essere l'ottavo di 15. Sarebbe interessante capire come e perché e come e perché quei risultati sono poi andati dispersi. Ho l'impressione che sia necessario uno sforzo straordinario - mi correggo - ordinario, cioè la creazione di condizioni ordinarie, le quali consentano di affrontare in modo efficace il problema della cosiddetta cosiddetta fase discendente, la trasposizione della normativa interna. Il motivo principale di questo ritardo è che il personale che presso un Ministero segue la trattativa con la quale si fa una direttiva non è lo stesso che che dopo cura la fase discendente ed i decreti legislativi. Abbiamo bisogno di vincolare il Governo all'istituzione presso ogni Ministero, di un nucleo di lavoro per le politiche

comincia a lavorare ai decreti legislativi. Come lo si può fare, non sapendo ancora come sarà fatta la legge comunitaria? Lo si può fare benissimo: se la legge comunitaria detterà particolari criteri di delega che interferiscono con il decreto legislativo, lo si potrà sempre correggere. Ma sarebbe bene che,

Questo richiede un cambiamento di mentalità, ma assicurerebbe la possibilità di fare tempestivamente i decreti legislativi

volte chi segue le trattative si batte fino al sangue per ottenere una virgola, un punto e virgola o due parole che consentano opportuni e prudenti adattamenti tesi a salvaguardare un settore produttivo italiano; se poi chi fa i decreti legislativi non è al corrente in dettaglio di come si è svolta la trattativa, perché è un'altra persona e non ha seguito la fase ascendente, è possibile, e spesso è accaduto,

politiche comunitarie, che segua sia la fase ascendente che quella discendente. Un problema ulteriore ricordato nell'ordine del giorno riguarda il modo con cui questi uffici vanno costituiti. Signor Ministro, non abbiamo personale adeguatamente preparato, e sa perché? Perché non facciamo uso dell'istituto degli esperti. Possiamo mandare alla Commissione gente che lavora con la Commissione e impara il diritto e le procedure, impara a conoscere le persone e si fa conoscere dalle persone.

Perché facciamo fatica a trovare candidati? Perché non abbiamo gli esperti. I francesi, i tedeschi e gli inglesi per ogni posto presentano tre, quattro,

qualità del nostro personale e a consentirci di costituire nuclei per gli affari comunitari di qualità, prepara il personale che poi possiamo inviare in quelle sedi per entrare negli alti livelli della burocrazia di Bruxelles. ciò richiede anche un'altra condizione: non si possono mandare come esperti quelli che danno fastidio e che si vuole allontanare dagli uffici romani. Bisogna mandare i migliori e, quando tornano, bisogna seguirli nel loro sviluppo professionale e di carriera, in modo da poter

Tutto ciò in spirito assolutamente *bipartisan,* con l'intento di aiutare ad affrontare, per una volta concretamente, un problema annoso su cui ho sentito fare molta retorica ma sul quale fino ad ora uno scambio di idee serio sulle ragioni

come Gruppo di Rifondazione Comunista-Sinistra Europea abbiamo condiviso in Commissione molti elementi presenti nella relazione e abbiamo votato favorevolmente, così come abbiamo giudicato in modo positivo alcuni emendamenti prodotti dalla discussione della Camera Peraltro, il nostro Gruppo parlamentare e il nostro partito si sentono fortemente coinvolti nella costruzione democratica dell'Europa, tanto che non a caso abbiamo voluto darci il nome di Rifondazione Comunista-Sinistra Europea, per indicare la dimensione dei nostri compiti e del nostro impegno. Interverrò soltanto su due elementi centrali, data la limitatezza della discussione. Tra poco, il 25 marzo 2007, a Berlino il Consiglio europeo avanzerà probabilmente una dichiarazione politica in relazione alla Costituzione europea e ai progetti costituzionali. È una discussione di grande ampiezza, che attiene esattamente al futuro della Comunità europea. La sconfitta del *referendum* in Francia e in Olanda non può essere considerata infatti un mero incidente di percorso, né tanto meno un irrazionale e retrogrado rifiuto nazionalista del progetto di unità del continente, ma attiene invece a due questioni di fondo, a due contraddizioni. La prima: ci siamo trovati di fronte alla natura elitaria e verticista della proposta di Costituzione, privata di un reale dibattito che coinvolgesse cittadine e cittadini. Ciò ha prodotto il disagio e la lontananza delle popolazioni: è un *vulnus* democratico a cui si deve porre rimedio. Le Costituzioni sono sempre il frutto di grandi discussioni, di battaglie politiche, di rivolgimenti e di partecipazione che ne hanno permesso proprio il loro carattere costituente: sono le modalità con cui si affermano i grandi cambiamenti sociali e politici. La rilevanza crescente delle decisioni operate su scala europea, per le implicazioni che hanno per l'intera popolazione del continente, impone un livello di legittimità democratica pari almeno a quella espressa negli Stati nazionali nel secondo dopoguerra. Per questo occorre una riapertura del dibattito sugli assetti costituzionali, che deve passare attraverso il coinvolgimento di tutte le istituzioni democratiche della società civile: un vero processo democratico e partecipato. Non serve una Costituzione concessa da un sovrano magnanimo, ma una vera partecipazione di popolo che possa riconoscersi in un comune destino e in un progetto sociale e politico. Ma dietro al rigetto di Francia e Olanda c'è un fenomeno ancor più complesso: c'è c'è il riflesso di una preoccupazione, anzi di una sofferenza per le politiche economiche e sociali prodotte nel corso degli ultimi due decenni, che si sono espresse sia nelle grandi scelte politico-economiche che nelle concrete direttive. Mi riferisco a quelle opzioni liberiste cristallizzate dal Trattato di Maastricht e dal Patto di stabilità che abbiamo criticato e che pensiamo siano alla base di stagnazioni e difficoltà economiche, ma anche alla base dei grandi rivolgimenti, della compressione forte su salari, occupazione, diritti sociali, condizioni di vita di milioni di persone e di una crescente precarietà per milioni e milioni di persone. È difficile considerare positiva una proposta costituzionale quando essa appare correlata a scelte economiche e sociali che mettono in discussione quel grado di stabilità e di diritti che fanno la differenza dell'Europa rispetto ad altre parti del mondo e che sono il frutto di 100 anni del movimento popolare e democratico e del movimento dei lavoratori e delle lavoratrici. Questo mi permette anche di esprimere qualche giudizio su un altro elemento di fondo della costruzione europea: la cosiddetta Strategia di Lisbona così come è stata definita nel 2000 e poi, poco poco più tardi, corretta nel Consiglio europeo del febbraio 2005. Da una parte, non possiamo che sostenere e condividere alcuni grandi obiettivi avanzati: conoscenza e innovazione per la crescita, Europa come luogo attraente per lavorare, piena occupazione e di qualità, centralità della ricerca e della conoscenza. Ma ci pare che questi obiettivi, altamente condivisibili, molte volte entrano in contraddizione con altri elementi proposti nella stessa Strategia di Lisbona e con il Patto di stabilità, tali da rendere i primi largamente impraticabili. Ci pare, ad esempio, difficile perseguire la buona occupazione e, nello stesso tempo, avere come stella polare la flessibilità del mercato del lavoro e una pratica generalizzata di rimessa in discussione di legislazioni garantiste del lavoro stesso, per non parlare della costante pressione per ridurre il costo del lavoro e la disarticolazione del sistema previdenziale pubblico. È difficile conciliare la formazione e la ricerca con la continua diminuzione della spesa pubblica; è difficile costruire un equilibrio produttivo su scala continentale, quando vi è una costante ricerca di riduzione del bilancio europeo e quando l'espressione «politiche industriali» sembra essere diventata tabù nel linguaggio e nelle pratiche politiche. A me pare che la strada che aveva fatto forte l'Europa, il suo sistema sociale, cioè la via dell'armonizzazione sia stata abbandonata da tempo per seguire la messa in concorrenza dei sistemi sociali. Per questo esprimo un particolare punto critico, già esternato in Commissione, sui processi di liberalizzazione, che molte volte (quasi sempre), significa privatizzazione e sulla cosiddetta direttiva Bolkestein, in discussione in questi giorni nel Parlamento europeo. Questa direttiva sui servizi punta ad organizzare la concorrenza diretta di lavoratori e lavoratici su scala europea, in piena contraddizione con la volontà conclamata di creare occupazione buona e stabile. di scelte che vanno in senso inverso a uno spazio europeo integrato ed armonizzato, che richiede invece servizi pubblici organizzati su scala europea. Essi sono beni di utilità collettiva, soddisfano bisogni elementari della popolazione e devono essere gestiti da strutture pubbliche (non automaticamente dallo Stato) per rispondere alla società e non alle esigenze di profitto. Se si deve inventare una cittadinanza europea, questa non può che essere definita sulla base dei diritti che garantisce, a partire dalla salute, da una vecchiaia serena, da un sistema articolato di sicurezze sociali e dalla scuola di qualità.

un'Europa che, senza tentare di rivaleggiare con le superpotenze, e senza lasciar loro campo libero, diventi il motore di un'altra mondializzazione, il suo stesso laboratorio». Occorre, usando le mie più semplici parole, un'Europa della democrazia, della libertà, della pace e della giustizia sociale.

di ciò che tutti auspicavamo e auspichiamo, pur da posizioni diverse (chi auspica l'Europa dei mercati, della libera circolazione delle persone

non vi è dubbio che questo processo di integrazione europea ha avuto una grave battuta d'arresto il 29 ottobre 2004, dopo che la città di Roma, come fu per il Mercato comune, ha avuto l'onore di essere sede della firma del Trattato per la Costituzione europea. Ricordo che allora ero già vice presidente della Commissione per le politiche europee, presieduta alla Camera da un parlamentare abbastanza vivace e intelligente, anche se con delle sue idee particolari, l'onorevole Stucchi, come ora ho l'onore di partecipare alla Commissione autorevolmente presieduta dal professore - mi piace chiamarlo così - Manzella,

Commissione senatoriale sulle politiche europee - gioimmo tutti anche perché eravamo in presenza (come auspico e i primi passi vanno in questo senso) di un Governo,

passi in avanti per essere pronta nel 2006 ad un Trattato costituzionale comune. Purtroppo - dirò anche i motivi che a mio parere sono alla base di questi no

piuttosto forte da Paesi terzi: un Paese che tende a chiudere le proprie frontiere, piuttosto che allargarsi in tema europeista (e parlo di un Paese retto da un Governo di centro-destra, che ha avuto i suoi drammi, come l'assassinio di Van Gogh ed altri). di Van Gogh ed altri). A mio avviso, la depressione che circondò questi due fatti si allargò poi ad altri Paesi. Non possiamo dimenticare che, subito dopo, la Gran Bretagna,

ha chiamato tutti a una pausa di riflessione che sarebbe stata ed è utile per capire cosa succede. Senatori Senatori della Repubblica, presidente e professore Manzella, ricordo che ci furono poi anche dei quesiti e qualcuno pensò a piani alternativi al Trattato costituzionale. Si pensò quindi che, se non era possibile rimettere in piedi il cammino di ratifica per i Trattati, sarebbe stato utile individuare percorsi alternativi. Su questo si innestò un momento importantissimo, quello avente ad oggetto l'eccezione del Governo britannico sulle politiche europee. Ricordo ai colleghi che io sono siciliano, sono stato parlamentare regionale nella mia Regione e anche uomo di Governo della Regione siciliana. Sappiamo quanto sia stato importante il contributo dell'Europa per risollevare le sorti economiche e infrastrutturali di alcuni Paesi.

un padre che meritò di entrare in Europa per i passi importanti da lui compiuti, come la visita in Israele, le posizioni europeiste, quegli agganci agli Stati Uniti d'America, non in posizione di vassallaggio, ma di fido alleato, che ancora oggi danno risultati importanti); ma la ragione fu fortemente economica, perché questi Paesi vedevano le loro economie incontrarsi. Non dimentichiamo che in Francia e Germania

malauguratamente, oltre ad altri aspetti. Ciò nonostante, la Turchia è riuscita a rimanere uno Stato laico che non ha subìto la malformazione dell'integralismo che altri Paesi malauguratamente, presidente Manzella, hanno subìto, in quell'area importante.

introduceva elementi inquietanti che ci avrebbero tra l'altro distanziato dagli altri *partner* europei. Con molta sapienza il presidente Manzella e la Commissione di merito hanno espunto un articolo che ci avrebbe impedito,

solida costruzione politica che sa difendere la pace nel mondo, non in vassallaggio e neanche in alternativa agli Stati Uniti, che rimangono un solido bastione di alleanza al quale questo Governo non può assolutamente, io spero, rinunciare.

anche se siamo d'accordo con molte delle valutazioni che sono state fatte e proposte anche dal Governo. Sono d'accordo, ad esempio, con chi sostiene che le radici dell'attuale crisi politica europea siano sostanzialmente di natura economica. Ciò investe, in particolar modo, le tre maggiori economie dell'Europa: Francia, Italia e Germania. Questi tre Paesi registrano, dall'inizio del decennio, tassi di crescita modesti: essi infatti mostrano gravi problemi di finanza pubblica che li ha portati a superare, negli ultimi anni e ripetutamente, i limiti di Maastricht, così come presentano situazioni difficili in tema di mercato del lavoro. Nel nostro Paese il tasso di disoccupazione è nettamente migliorato, scendendo al 7,7 per cento, grazie soprattutto all'azione prodotta dalla riforma del mercato del lavoro, anche conosciuta come legge Biagi, fortemente voluta dal Governo Berlusconi in omaggio a quella strategia di Lisbona nella quale si incardina ogni intervento europeo per la crescita e lo sviluppo. È un'Europa che si è dato l'ambizioso obiettivo di fare dell'Unione, entro il 2010, l'economia più dinamica del mondo basata sulla conoscenza e il nostro Paese ha svolto fra le migliori *performance* nella creazione di posti di lavoro, secondo solo alla Spagna, nonostante un livello di crescita - il nostro - decisamente inferiore. Guai a noi se oggi interrompessimo questo processo, tornando indietro rispetto all'ottima legge Biagi, assecondando una cultura veterocomunista che pensa che il lavoro e i posti di lavoro si creino per decreto-legge. Non potrà esserci condivisione da parte nostra di nessun PICO (il piano per l'innovazione, la crescita e l'occupazione), se il piano italiano, quando il Governo con la finanziaria del 2007 lo cofinanzierà, non salvaguarderà lo spirito della legge Biagi e del pacchetto Treu, al quale riconosciamo di aver avviato con grande coraggio e difficoltà nel nostro Paese la riforma del mercato del lavoro, modernizzando un sistema arcaico, tutto ispirato a un pansindacalismo che ancora avvolge l'Aula di questo ramo Abbiamo la necessità di prendere atto del fatto che la flessibilità guidata del mercato, salvaguardata da un sistema di regole giuste, non è più un obiettivo che possiamo tralasciare e non è più una scelta facoltativa: è una necessaria scelta da parte di tutti. Guai a noi se continuassimo quindi a dividerci in modo sterile tra fautori e oppositori delle riforme strutturali che l'Europa ci chiede e che attengono alle competenze di politica economica ancora in capo agli Stati nazionali, e se ci occupassimo pochissimo di ampliare il mercato interno, cruciale competenza comunitaria alla quale vogliamo concorrere. Merci e capitali si muovono liberamente, sono in gran parte rimossi gli ostacoli alla libera circolazione delle persone, anche se barriere invisibili, come le differenze linguistiche e culturali, permangono ed incidono sulla libertà dei prestatori di servizi e quindi sulla libera circolazione dei servizi. E poiché oggi i servizi rappresentano più del 70 per cento dell'occupazione e del reddito dell'Unione, il mercato interno dei servizi è il settore più importante per il rilancio dell'economia europea. All'articolo 10 di questo disegno di legge abbiamo avuto l'opportunità, grazie all'iniziativa dei senatori Girfatti e Silvestri e alla condivisione del ministro Bonino, di dimostrare che al Governo italiano, al Parlamento italiano sta a cuore tanto il lavoro degli italiani quanto la libertà dei servizi. Nonostante l'impostazione del vice ministro Pinza, che mirava a cancellare per decreto la figura professionale del consulente finanziario, l'attenzione e la sensibilità di coloro che ho citato, che hanno avuto a cuore, oltre al lavoro, anche la reale tutela del risparmiatore in Italia, si è potuta eliminare un'ingiustizia, consentendo al professionista di continuare ad esercitare la sua professione e a crescere, in un quadro europeo che lo vuole libero di circolare tra gli Stati membri e possibilmente libero da conflitti di interessi, poiché l'unico interesse del quale si fa carico è quello del risparmiatore. L'assenza di conflitti di interessi è l'elemento cardine che distingue questa figura dagli altri operatori del settore, come le banche o le società per azioni, e permette al professionista di non essere influenzato dalle commissioni pagate dagli intermediari. È importante sottolineare che nei Paesi finanziariamente più evoluti, dove è ben radicata, la figura del consulente finanziario indipendente, ha contribuito ad una maggiore efficienza del mercato, con la conseguente riduzione dei costi per i risparmiatori, una migliore gestione dei rischi e la protezione del patrimonio dagli scandali finanziari. Ecco perché il rischio operativo del consulente è nullo ed è per questo motivo che la direttiva prevede per il consulente la sola sottoscrizione di una polizza assicurativa professionale, come per tutti i liberi professionisti, oltre ai requisiti di professionalità e onorabilità. Infatti, la Commissione bilancio, nella cui deliberazione ci ritroviamo, ritiene opportuno prevedere che l'esercizio nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento sia reso possibile, limitatamente al mero servizio di consulenza in materia di investimenti, alle persone fisiche in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB. Ecco, signora ministro Bonino, questa è l'Europa che noi di Forza Italia desideriamo costruire e le cui direttive volentieri riceviamo, e che possiamo sostenere soprattutto se concorriamo a scriverle, come ci ha ricordato molto bene prima il senatore Buttiglione. Noi aderiamo a un'idea di Europa sempre più attenta a coniugare lo sviluppo, i diritti, l'identità e la libertà, che in questa legge comunitaria non ritroviamo per interi. Forza Italia, attraverso la nostra dichiarazione di voto finale, spiegherà qual è l'Europa che invece vogliamo contribuire a costruire.

ovvero all'introduzione di un meccanismo di contribuzione diretta dei cittadini al bilancio dell'Unione Europea, anche per rafforzare il rapporto, appunto tra i cittadini e l'Unione,

dei controlli. Com'é noto, vi è un controllo esercitato dalla Corte dei conti europea, in collaborazione con la Corte dei conti degli Stati membri, e vi è un controllo esercitato dal soggetto responsabile dell'attuazione del bilancio, cioè la Commissione europea, che riferisce annualmente al Parlamento europeo.

degli Stati membri nella definizione delle procedure di controllo della spesa comunitaria e chiedendo, poi, agli Stati membri di rilasciare annualmente una dichiarazione di affidabilità della spesa, ovvero di efficacia e di legalità nelle procedure di spesa. Gran parte dei Paesi hanno già definito o stanno definendo procedure che collocano quest'attività di controllo a livello di Governo e dei Parlamenti nazionali, in tal modo unificando i controlli che vengono effettuati dai vari centri di spesa, dai vari organismi erogatori della spesa. Ma l'Italia non ha ancora avviato, come il Ministro sa bene,

questo tema di particolare rilievo. Vorremmo cioè che il Governo si impegnasse ad attivare tutte le iniziative iniziative volte ad individuare gli strumenti di coordinamento dei controlli, oggi diversificati e ricadenti su molteplici centri di spesa e autorità, anche locali, e a fare in modo che ci si possa presentare in sede comunitaria con una procedura, speriamo nei prossimi mesi, definita, tale da consentire al Governo stesso, al Ministero dell'economia, ma anche al Parlamento, di partecipare al controllo e di cooperare alla definizione della procedura in sede comunitaria.

devo ringraziare preliminarmente quei colleghi che si sono resi solidali per la ristrettezza in cui questa discussione è stata costretta. Peraltro, è stata una discussione di stampo europeo, perché in poco tempo abbiamo toccato dei temi fondamentali per l'Europa e per la partecipazione dell'Italia nell'Unione Europea. Mi riferisco, ed esprimo contestualmente parere favorevole, all'ordine del giorno G104, presentato dai

Silvestri, in materia di Erasmus. Proprio oggi un grande quotidiano europeo metteva in luce come l'Erasmus sia uno dei meccanismi più fecondi nella dinamica dell'Unione Europea.

senatori, che ha introdotto la grande suggestione delle piante che scompaiono; una suggestione antimercantilista che non possiamo non condividere.

ha introdotto il tema dello specifico sociale europeo, ricordando come il 25 marzo prossimo saremo tutti chiamati ad un appuntamento di Il senatore Girfatti ha messo in luce gli emendamenti migliorativi introdotti in Commissione. Il senatore Strano ha svolto un'analisi sul momento momento costituzionale europeo e sulla particolare posizione dell'Italia in questo - speriamo - risveglio costituzionale che ci sarà con la presidenza tedesca. Infine, l'intervento della senatrice Bonfrisco ha il tema della Strategia di Lisbona e della libertà di circolazione dei servizi: due temi fondamentali che certo in questa sede non si è potuto non si è potuto approfondire sino alle ultime conseguenze, ma che sono stati - per così dire - semi gettati per il prossimo lavoro in Commissione e in Assemblea.

condenso in un auspicio il senso di un'eco del dibattito, che, per quanto siano stati contenuti i tempi, è stato tuttavia intenso e svolto con unanime passione europea. Esprimo l'auspicio che la prossima relazione annuale, che tra l'altro vedremo tra pochissimi mesi, possa segnare per l'Italia una fase di rilancio e di sviluppo del progetto dell'Unione.

Mi riferisco, per esempio, agli interventi del senatore Eufemi, del collega Buttiglione, così come di molti che sono intervenuti su punti specifici. Quindi, esprimerò la mia valutazione uno per uno sugli ordini del giorno.

essere europeisti significa approvare questa legge comunitaria al massimo entro domani mattina, procedere velocemente anche alla Camera e, per favore, girare pagina, cominciare da capo. Lo dico con grande rispetto al collega Selva: abbiamo bisogno, semmai, di un grande dibattito, con mozioni, sull'Europa, sul Trattato, su come organizzare. Credo che oggi concretamente il segnale più serio che possiamo dare è approvare legge comunitaria al massimo domani, consentire un passaggio forse alla Camera, ma finalmente girare pagina. Quindi, mi riservo in altre sedi dibattiti sull'Europa. Il Governo accetta tutti gli ordini del giorno come raccomandazione. Uno per uno posso fornire anche elementi di spiegazione, dalle sementi all'organizzazione. Caro collega Buttiglione, capisco lo spirito di aiuto, ma capisco anche che quello di così necessario scritto nel suo ordine del giorno ha implicazioni finanziarie e comporta una ristrutturazione anche delle carriere dei funzionari. il Governo lo accetta come raccomandazione, essendo inteso che questi cambiamenti, se non sono stati fatti negli ultimi dieci anni, ci sarà anche un motivo di vera e propria difficoltà, con tutta evidenza. Il nostro impegno dev'essere di una rapida una rapida nuova legge comunitaria già all'inizio dell'anno prossimo e credo anche, però, di un dibattito politico sull'Europa e il rapporto Italia-Europa. Questo credo sia indispensabile, in particolare alla vigilia del 25 marzo e quindi del cinquantenario della firma del

Quindi, votiamo gli ordini del giorno, vediamo a che ora arriviamo, tenendo conto che ci sono state varie richieste, considerando anche il fatto che alle ore 21 sono convocate la Commissione bilancio e la Commissione finanze, quindi c'è ancora un lavoro intenso da fare.

PRESIDENTE. Siamo di fronte al fatto che la Commissione ha espresso un'opinione favorevole, il Governo l'accetta come raccomandazione. Credo che forse si può ricostruire il tessuto unitario dicendo ai presentatori che c'è un accoglimento di massima degli ordini del giorno, che mi pare anche questo significativo, senza che si vadano a votarli, che non mi sembra francamente una condizione.

che impatta su molti elementi di bilancio, mi è sembrato già utile dire che il Governo lo accetta come raccomandazione.

a livello internazionale e nazionale. È una questione economica di rilievo e vorrei comprendere per quale motivo, al contrario di quanto detto dal relatore,

Il Governo conosce quanto lei, senatrice De Petris, gli articoli 5 e 6 del Trattato, e conosce sicuramente quanto lei le implicazioni e l'importanza della tutela delle sementi. Non è l'unica, mi creda, senatrice.

dichiarato di avere in elaborazione una seconda direttiva comunitaria al riguardo, il Governo, credo prudentemente e responsabilmente, ritiene di accogliere l'ordine del giorno G103 come raccomandazione. Le preoccupazioni sono le stesse, le procedure sono un po' diverse.

Sono consapevole del fatto, signor Ministro, che l'ordine del giorno comporta qualche costo per lo Stato. Questa è la ragione per la quale abbiamo formulato un ordine del giorno e non un emendamento, che in questa fase sarebbe stato assai difficilmente realizzabile. La invito, però, ad avere fiducia: le resistenze della macchina burocratica possono essere spezzate.

che questo divenga un emendamento da proporre all'unanimità per la prossima legge comunitaria, nel caso che il Governo non provveda tempestivamente a dargli esecuzione. Per il momento, va bene che venga accolto come raccomandazione, ma non è che si accoglie la raccomandazione perché un ordine del giorno, come un sigaro, non si nega a nessuno:

nuova finestra"), *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sul testo. Esprime altresì parere non ostativo sugli emendamenti, ad eccezione delle proposte 15.0.2, 15.0.3, 15.0.4 e 23.2 sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione». «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 15.0.4 (testo 2), trasmesso dall'Assemblea e relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo».

La seduta è tolta